L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure

lungo e difficile, che abbiamo da poco messo alle nostre spalle, ho costantemente informato il Parlamento, relazionando, sia in Aula che nelle Commissioni competenti, sull'andamento della pandemia e relativamente alle misure che il Governo ha adottato per contrastare una diffusione incontrollata del virus, che ha stravolto le nostre vite. Come ho più volte ripetuto negli ultimi mesi, non considero questo appuntamento un atto dovuto, da svolgere semplicemente in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 il lavoro del Parlamento e la leale collaborazione tra Governo, Regioni, Province autonome e Comuni che in tutti i passaggi più difficili ci hanno consentito di resistere e tenere coeso il Paese, anche quando siamo stati investiti dalle onde più alte di questa emergenza sanitaria senza precedenti. Dal 20 febbraio, dai primi casi di Codogno, è stato subito chiaro a tutte le persone responsabili e di buona volontà che, senza uno sforzo unitario delle istituzioni repubblicane e di ogni cittadino, non si sarebbe arginato, né tantomeno sconfitto, questo nemico incredibilmente forte che, all'improvviso, ci ha costretto a rinunciare a libertà personali, che ritenevamo inattaccabili, e ha colpito duramente le nostre attività economiche e sociali. Non c'è altra strada diversa dall'unità per affrontare l'emergenza sanitaria, economica e civile più grande che abbiamo conosciuto dal Dopoguerra. Sono state illuminanti, a tal proposito, le parole del presidente Mattarella, a cui va la nostra gratitudine, nel suo discorso alla Nazione di fine anno. *(Applausi)*. con la preoccupazione che vivo da Ministro della salute, anche rispetto alle tensioni di questi giorni, voglio rivolgere a tutti un accorato messaggio di responsabilità, per l'unità a Roma, come in tutte le Regioni della nostra Italia. Mi rivolgo con lo stesso spirito alla maggioranza e all'opposizione: siamo nell'ultimo miglio, a un passaggio delicato e decisivo, per vincere finalmente la lunga e difficile battaglia che stiamo conducendo da mesi contro un terribile nemico invisibile. Adesso, ancor di più che in altre fasi dell'emergenza, serve uno sforzo unitario, una leale collaborazione, a Roma come in tutte le Regioni. Le prossime settimane e i mesi che verranno saranno difficilissimi, perché il virus può tornare a colpirci duramente e perché dovremo contemporaneamente portare avanti la più grande campagna di vaccinazione della storia recente. Sarà tutto terribilmente complicato. Ecco perché insisto: nei prossimi giorni teniamo fuori e lontana dalla battaglia politica, da vere o presunte tensioni elettorali, la salute degli italiani. Sarebbe davvero un errore imperdonabile distrarci o rallentare a poche centinaia di metri dal traguardo. Una forte e leale collaborazione istituzionale, un Paese intero che si stringe a coorte è certamente anche la via maestra per essere vicini ai nostri medici, infermieri, personale sanitario, che ogni giorno da mesi combattono in prima linea e che in queste ore sono impegnati in modo straordinario anche nella campagna di vaccinazione. Dobbiamo ringraziarli tutti ed essere uniti e coerenti nel sostegno al Servizio sanitario nazionale è anche il modo più concreto per valorizzare il lavoro prezioso e insostituibile che essi svolgono. Con l'avvio della campagna di vaccinazione - come è stato detto più volte in queste giornate - finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel che stiamo attraversando. Adesso sappiamo con ragionevole fiducia che il Covid ha i mesi contati e che, grazie a uno sforzo senza precedenti della comunità scientifica, con i nuovi vaccini sconfiggeremo anche questo virus che ha colpito così duramente il nostro Paese. Mi sia consentito di rimarcare il ruolo della scienza dentro questa partita: la conoscenza, la ricerca, la capacità delle migliori intelligenze di lavorare insieme hanno prodotto questo risultato straordinario. Mai nella storia un vaccino era stato così veloce: dobbiamo ricordarlo sempre, soprattutto quando decidiamo dove investire le risorse pubbliche. La scienza sta illuminando la strada che ci porterà fuori da una stagione terribile e noi dobbiamo investire, ogni giorno di più, sui nostri ricercatori che ringraziamo e di cui siamo orgogliosi. È vero: finalmente vediamo la luce e possiamo affrontare con più fiducia i prossimi mesi, ma non abbiamo ancora vinto. Facciamo molta attenzione e non sbagliamo la lettura di questa fase decisiva. La nottata non è ancora passata: l'ultimo miglio è ancora lungo e irto di ostacoli da superare. Dobbiamo affrontarlo con rinnovata fiducia, ma senza abbassare la guardia e tenendo saldamente i piedi per terra. Certo, siamo tutti felici e orgogliosi per l'avvio della campagna nazionale di vaccinazione, per i primi incoraggianti risultati raggiunti, ma siamo solo all'inizio, alle prime battute di una lunga e difficile maratona. Ma soprattutto - questo è il punto che mi preme mettere subito in evidenza dovremo continuare a convivere con una forte circolazione del virus sino a quando le vaccinazioni non avranno un positivo effetto epidemiologico. Lo dico con chiarezza e con il senso di responsabilità che sento nei confronti del Paese, con parole semplici e spero chiare: attenzione, in tutta Europa sta montando nuovamente una forte tempesta. Angela Merkel ha detto la verità quando ha affermato che ci aspettano i mesi più duri della pandemia. Il virus, quando verranno autorizzati e poi distribuiti ulteriori vaccini, verrà piegato, ma adesso continua a circolare con forza crescente e può di nuovo colpirci molto duramente. Non dobbiamo farci alcuna illusione: i prossimi mesi saranno difficili e, se li affrontiamo pensando che siamo già fuori pericolo, andiamo incontro a drammatiche disillusioni. Nell'anno che è alle nostre spalle abbiamo, purtroppo, imparato che i numeri, nella loro progressione e connessione, sono come il barometro che, con la bassa pressione, anticipa l'arrivo di una nuova tempesta. Nel mondo i numeri restano terribili nella loro evidente drammaticità: un caso confermato ogni 89 abitanti e un decesso ogni 4.080 abitanti. Sono numeri impressionanti che, ancora una volta, si commentano da soli. In Europa, purtroppo, attualmente la situazione è peggiore: un caso confermato ogni 27 abitanti e un decesso ogni 793 abitanti. Mentre si svolge questo nostro dibattito, grandi Nazioni come la Germania e il Regno Unito sono in *lockdown* totale. La Gran Bretagna è al terzo *lockdown* dalla scorsa primavera, questa volta anche con le scuole chiuse. La Germania ha per la prima volta superato per più giorni di fila i 1.000 decessi al giorno; l'Inghilterra sfonda il numero dei 60.000 casi quotidiani, la Francia è vicina a 3 milioni di contagiati e continua ad avere circa 20.000 nuovi casi ogni ventiquattr'ore ore; la Spagna, all'8 gennaio, ne ha registrati 25.000 per la prima volta anche la Svezia, che non ha mai adottato severe misure restrittive di contenimento, si è dotata di una legge nazionale che conferisce al Governo il potere di decidere *lockdown* totali. In questo contesto europeo pesano anche le valutazioni sulla maggiore capacità di trasmissione delle varianti del virus, a partire da quella diffusa in Gran Bretagna, che i nostri scienziati stanno approfondendo anche grazie al lavoro di sequenziamento che è stato molto rafforzato nelle ultime settimane. In Italia non facciamoci portare fuori pista dalla circostanza che attualmente abbiamo un numero di casi leggermente più basso rispetto ad alcuni altri grandi Paesi europei. I dati dell'ultima cabina di monitoraggio sono molto chiari e non vanno assolutamente sottovalutati. Questa settimana si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese: aumentano contemporaneamente RT, incidenza, tasso di occupazione delle terapie intensive e i focolai di origine sconosciuta. Per essere ancora più preciso, riporto, anche se in modo schematico, i principali dati emersi dall'ultima cabina di monitoraggio. Partiamo dall'RT: 15 e il 28 dicembre 2020, dopo quattro settimane torna a crescere l'RT e per la prima volta, dopo sei settimane, è ora sopra l'indice 1. Già questo dato, preso singolarmente, indica chiaramente che siamo molto probabilmente a un nuovo cambio di fase: l'epidemia è di nuovo in una fase espansiva. I dati ci dicono che l'RT calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,03; 3 Regioni hanno un RT puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore; 6 Regioni lo superano nel valore medio; una Regione lo raggiunge e 3 lo sfiorano. L'incidenza nazionale a quattordici giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita. Negli ultimi quattordici giorni passiamo da 305,47 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo tra il 14 e a 313,28 casi nell'arco temporale che va dal 21 dicembre al 3 gennaio. Nonostante la settimana in valutazione sia stata caratterizzata da un numero più basso di tamponi nelle giornate festive, si osserva di nuovo un aumento dell'incidenza, che nel Paese è oggi pari a 166,02 per 100.000 abitanti in una settimana. Come rileva il *report* della cabina di monitoraggio, l'incidenza su tutto il territorio è dunque ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e del tracciamento dei contatti. Con un valore di incidenza settimanale pari a 166, siamo a un dato 3 volte maggiore del tetto di 50 nuovi casi, considerata la soglia massima gestibile dai servizi sanitari territoriali. Non c'è da meravigliarsi, quindi, se aumenta sensibilmente il numero di nuovi casi non riconducibili a catene di trasmissioni note, passati da 31.825 a 40.487. L'altro effetto automatico dell'aumento del tasso di incidenza è il progressivo sovraccarico delle strutture ospedaliere. Sempre dal *report* della cabina di monitoraggio si rileva che sono passate da 10 a 13 le Regioni e le Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e in area medica sopra la soglia critica. In particolare, per quel che riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive, va rilevato che, a livello nazionale, esso torna ad attestarsi sopra la soglia critica del 30 Dai parametri precedentemente riportati consegue un mutamento significativo dell'indice di rischio attribuito alle singole Regioni: dodici Regioni e Province autonome sono ad alto rischio;

peggiorano contemporaneamente, abbiamo l'obbligo di prendere nuove misure, proporzionali al rischio di una diffusione incontrollata dell'epidemia. Per le ragioni che ho finora esposto, il Governo ritiene inevitabile prima di tutto prorogare al 30 aprile lo stato di emergenza che scade il 31 di gennaio. Questo passaggio, ampiamente giustificato da tutte le argomentazioni epidemiologiche finora riportate, consente all'architettura istituzionale dell'emergenza, impegnata in queste ore anche nella campagna di vaccinazione, di continuare a esercitare le sue funzioni e il suo fondamentale lavoro. Nella giornata di lunedì, attraverso un confronto con le Regioni, abbiamo avviato anche il lavoro per la stesura del nuovo DPCM, che sostituirà quello in scadenza il 15 di gennaio. Nel nuovo decreto prevediamo una conferma delle misure fondamentali già vigenti e del modello per fasce differenziate, che ci ha consentito di abbassare la curva tra novembre e dicembre. È inoltre intenzione del Governo confermare il divieto di spostamenti tra Regioni anche in zona gialla; ridurre gli assembramenti negli spazi antistanti i locali pubblici a rischio di aggregazione (attraverso il divieto di asporto per i bar a partire dalle ore 18); confermare l'indicazione di poter ricevere a casa massimo due persone non conviventi, come già avvenuto durante le vacanze di Natale, e stabilire l'ingresso in area arancione di tutte le Regioni a rischio alto, secondo i 21 parametri definiti dal decreto ministeriale del 30 aprile. È inoltre intenzione del Governo stabilire una quarta area, oltre a quelle rosse, arancioni e gialle: un'area bianca, che potrà scattare solo con livelli epidemiologici molto bassi (incidenza sotto i 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, RT sotto 1 e indice di rischio basso). In questa area le limitazioni saranno relative alle regole fondamentali del distanziamento e dell'utilizzo delle mascherine. È difficile che questa area possa scattare a breve, ma iniziamo a indicare un percorso di speranza per i mesi a venire. Con lo stesso spirito è intenzione del Governo, in area gialla e sempre nel pieno rispetto di tutte le misure di distanziamento, riaprire i musei come luogo simbolico della cultura del nostro Paese. Voglio venire ora alla seconda parte della mia relazione, quella relativa ai vaccini, e voglio ricordare in premessa che il 2 dicembre ho illustrato, sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei deputati, il Piano strategico nazionale di vaccinazione, con voto finale sulle mie comunicazioni. Il nostro è stato il primo Parlamento europeo a discutere e ad assumere il documento di indirizzo e programmazione per la somministrazione dei vaccini. Successivamente, il 17 dicembre c'è stato un passaggio formale in Conferenza Stato-Regioni.

È grazie a questo lavoro preparatorio, partito con largo anticipo anche rispetto al passaggio parlamentare, che il nostro Paese si è fatto trovare pronto, nonostante l'EMA abbia autorizzato il primo vaccino di Pfizer BioNTech circa un mese prima di quanto inizialmente previsto. previsto. A ieri notte abbiamo somministrato circa 800.000 dosi: un buon risultato, che attualmente ci fa essere la Nazione dell'Unione europea che ha somministrato il maggior numero di vaccini. Non rincorriamo le classifiche, ma credo che sia una soddisfazione per tutti vedere che oggi noi siamo i primi in quella graduatoria. Ecco perché voglio ringraziare il commissario straordinario per l'emergenza; voglio ringraziare la sua struttura, tutte le Regioni, le Province autonome e il ministro Boccia per il loro prezioso lavoro; il ministro Guerini per l'importante collaborazione delle nostre Forze armate; l'Aifa, l'Agenas, l'Istituto superiore di sanità, il Consiglio superiore di sanità e, naturalmente, il personale del Ministero della salute che, da mesi, è sotto una pressione senza precedenti. Quel che mi preme innanzitutto è mettere in evidenza il proficuo gioco di squadra che stiamo riuscendo a mettere in campo e che rappresenta - com'è del tutto evidente - la precondizione indispensabile per il successo della nostra iniziativa. Dobbiamo andare avanti così. Ci vogliono piena e totale collaborazione istituzionale, zero polemiche e un grande lavoro comune assicurato da un costante e puntuale lavoro di coordinamento nazionale. Voglio ripeterle ancora una volta che siamo solo all'inizio del nostro lavoro di vaccinazione: questa campagna, che per dimensioni non ha eguali nella storia recente delle Nazioni, è una lunga e difficile maratona, non una gara di velocità. Ecco perché guardiamo con soddisfazione alle attuali statistiche, ma siamo tutti consapevoli che siamo solo all'inizio e che c'è ancora tantissimo da fare per raggiungere nuovi risultati e portare avanti il nostro lavoro. Possiamo e dobbiamo farlo avendo chiari obiettivi, tempi e strategia per raggiungere i risultati attesi. Al Parlamento e a tutti gli italiani voglio trasferire un messaggio di fiducia: l'Italia, il Governo nazionale, le Regioni, le Province autonome e il Servizio sanitario nazionale sono pronti ad aumentare notevolmente il numero di vaccinazioni da effettuare quotidianamente appena saranno autorizzati nuovi vaccini. L'Italia è un grande Paese assolutamente in grado di garantire un numero di vaccinazioni adeguato al nostro fabbisogno. Per raggiungere questo obiettivo servono una grande organizzazione, un esercito di vaccinatori e, soprattutto, il clima giusto.

Lo dico con lo stesso spirito alle forze politiche che in quest'Aula sono opposizione e alle forze di maggioranza che sono, invece, all'opposizione nella maggioranza delle Regioni del nostro Paese. È troppo importante l'obiettivo che perseguiamo per macchiarlo con polemiche inutili che fanno male a tutti e, in particolare, agli italiani che, con il vaccino, possono e devono uscire da questo lungo incubo che noi tutti stiamo vivendo. Unità, unità, unità sulla campagna nazionale di vaccinazione. Il pieno successo della campagna di vaccinazione è di tutto il nostro Paese e non di una parte politica. Ecco perché non dobbiamo alimentare polemiche autolesioniste anche per il prestigio del nostro Paese. Oggi il vero problema a livello globale è la scarsità dei vaccini a disposizione rispetto alla fortissima domanda mondiale. Non ci sono scorte accumulate e dimenticate in qualche magazzino e non ci sono produttori di vaccino in qualsiasi parte del mondo che dispongano di fiale regolarmente autorizzate alle quali colpevolmente non ci si rivolge per acquistarle. L'Italia è stata la prima, con la Germania, la Francia e l'Olanda, a lanciare l'alleanza per i vaccini e a promuovere poi la decisione di affidare alla Commissione europea e non ai singoli Stati nazionali il ruolo di opzionare prima e acquistare dopo tutti i vaccini che con studi clinici attendibili fossero in una fase avanzata di sperimentazione. Ribadisco la nostra convinzione: il vaccino è un bene pubblico globale, diritto di tutti e non privilegio di pochi. Per questo in Italia esso è gratuito e gli acquisti sono effettuati direttamente dallo Stato, che lo distribuisce alle Regioni. A oggi abbiamo siglato opzioni per circa 226 milioni di dosi, che nelle prossime settimane aumenteranno ulteriormente fino a giungere circa 250 milioni, esercitando sempre il diritto di opzione previsto dagli accordi europei che ci consente di bloccare per ogni contratto siglato dall'Unione il 13,46 per cento dei vaccini. Così facendo abbiamo opzionato quasi il doppio delle fiale necessarie per vaccinare tutti gli italiani. Tutto quello che si poteva e doveva fare per approvvigionarsi del vaccino è stato fatto con attenzione e per tempo, muovendoci sempre guidati dal principio di massima precauzione. Adesso non possiamo far altro che continuare a utilizzare presto e bene le dosi di cui disponiamo; attendere con fiducia l'autorizzazione di nuovi vaccini e continuare a curare ogni singolo dettaglio per essere pronti ad accelerare quando avremo molti più vaccini a disposizione. Tutti noi, in Italia e in Europa, siamo ragionevolmente fiduciosi che l'aumento delle dosi disponibili avverrà in tempi non lunghi. La ricerca scientifica negli ultimi mesi ha compiuto un lavoro straordinario, senza precedenti nella storia mondiale.

Tutti, nel mondo e in Europa, vogliamo correre nella campagna di vaccinazione. Tutti non vediamo l'ora di riconquistare le libertà perdute e di far ripartire la nostra società e le nostre economie. Tutti sappiamo quanto siano decisivi i vaccini. Tutti, anche in Italia, vogliamo correre, ma dobbiamo farlo in assoluta sicurezza e con la massima trasparenza. Ecco perché è indispensabile dare agli scienziati e all'EMA tutto il tempo necessario per completare il loro lavoro. Solo così possiamo essere certi che, quando un vaccino è autorizzato all'immissione in commercio, esso è davvero efficace e sicuro. Fare presto e bene è possibile e io credo che non trascorreranno troppe settimane prima che venga autorizzato anche il terzo vaccino. A proposito della quantità di dosi a disposizione dell'Italia, voglio aggiornare il Parlamento rispetto alla mia precedente informativa del 2 dicembre. Ad oggi solo due vaccini sono stati autorizzati da EMA; il primo, Pfizer BioNTech, il 23 dicembre; il secondo, quello di Moderna, il 6 gennaio. Riceviamo per il primo trimestre da Pfizer 470.000 dosi a settimana e da Moderna 1.300.000 dosi in tutto il primo trimestre. Sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, l'EMA può procedere all'autorizzazione del terzo vaccino a partire dalla fine di gennaio. Una data segnata in rosso sul calendario è quella del 29 di gennaio. Con il vaccino AstraZeneca avremo a disposizione altre dosi fondamentali per la nostra campagna di vaccinazione. Sempre nel primo trimestre dell'anno è attesa l'autorizzazione anche per il vaccino Johnson & Johnson. Aggiungo sulle forniture un'ulteriore informazione: negli ultimi giorni la Commissione europea ha annunciato l'acquisto di altre 300 milioni di dosi Pfizer BioNTech per un'ulteriore fornitura di vaccini che, per l'Italia, significherebbe altre 40 milioni di dosi, di cui le prime 9 a disposizione già dal secondo trimestre. Altre interlocuzioni sono in corso con Moderna, che ha già aumentato le proprie forniture all'Europa da 80 a 160 milioni di dosi, di cui 20 destinate al nostro Paese. Voglio inoltre ricordare con particolare piacere il vaccino Reithera che è sostanzialmente tutto italiano e i cui risultati di fase 1 sono molto incoraggianti. Credo risulti chiaro a tutti in quest'Aula che è stato dispiegato un lavoro a tutto campo per approvvigionare l'Europa e, dunque, anche l'Italia, dei vaccini necessari per sconfiggere definitivamente il Covid nei tempi più brevi possibili. Con la stessa attenzione e determinazione stiamo lavorando parallelamente a organizzare nel dettaglio le forze che ci serviranno per portare avanti la campagna di vaccinazione, quando il numero di fiale disponibili aumenterà sensibilmente. L'Italia è pronta a mettere in campo una squadra forte e larga. Alle migliaia di personale che già lavorano in questi giorni nelle Regioni si aggiungeranno gli oltre 40.000 medici di medicina generale; i circa 7.500 pediatri di libera scelta; i potenziali 15.000 professionisti reclutati con il bando del commissario straordinario all'emergenza. Sono donne e uomini del Servizio sanitario nazionale; in tutte le Regioni, dalle grandi città al più piccolo Comune della nostra Italia, dopo aver combattuto ogni giorno per un anno, saranno ancora in campo per la sfida più importante, quella decisiva della campagna di vaccinazione. A tutti loro voglio rivolgere un doppio ringraziamento: grazie per quello che avete fatto in questo anno e grazie per quello che continuerete a fare nei prossimi mesi con il vostro lavoro prezioso ed insostituibile. In questo importante lavoro, come già deciso dal Parlamento, saranno impegnate anche le nostre farmacie, che potranno mettere a disposizione spazi e professionalità capaci di rafforzare la nostra offerta vaccinale. In sintonia con il piano nazionale vaccini, le prime tappe della nostra campagna di vaccinazione sono chiare e definite: innanzitutto il personale sanitario, le RSA e gli italiani dagli ottant'anni in su. Si tratta di oltre 6 milioni di persone, di cui più di 4 milioni sono gli italiani sopra gli ottant'anni. Al termine di questa prima e seconda fase avremo raggiunto tre obiettivi molto importanti: il primo, mettere in sicurezza il nostro personale sanitario, che ha pagato un prezzo altissimo anche in termini di vite umane e che è la nostra prima linea di questa battaglia; il secondo, mettere in sicurezza i nostri ospedali e le RSA; il terzo, difendere i nostri anziani, che sono stati i più duramente colpiti, in termini di perdita di vite umane, dal diffondersi di questa pandemia. Sono scelte che, insieme alle misure che adotteremo per contrastare una forte diffusione del contagio, potranno finalmente abbassare in maniera sensibile il numero di uomini e donne che ogni giorno in Italia perdono la vita in seguito al contagio da Covid. Aver scelto questa priorità nella campagna di vaccinazione rappresenta un tratto di umanità e di civiltà che credo sia profondamente giusto. Non credo ci possano essere dubbi: il Servizio sanitario nazionale, tanto più in una grave emergenza sanitaria, ha l'obbligo di tutelare innanzitutto il diritto alla salute, a partire dai più deboli, da coloro che corrono più rischi di perdere la vita. Credo che insieme possiamo fare un buon lavoro e raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Ci sono le condizioni per farlo. Ero e resto convinto che in un clima positivo e di dialogo la stragrande maggioranza degli italiani deciderà di vaccinarsi senza necessità di ricorrere all'obbligo. A chi ha dubbi dobbiamo rispondere con la trasparenza, con la trasparenza, con l'evidenza scientifica, con la capacità di ascolto e di dialogo *(Applausi)*, non con gli insulti, non con una guerra ideologica tra *fan* della scienza e primitivi delle caverne. Detto ciò, non vi è alcun dubbio che per il Governo resta fondamentale l'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge, che perseguiremo con ogni energia. Come recita l'articolo 54 della nostra Costituzione, chi svolge funzioni pubbliche ha il dovere di farlo «con disciplina ed onore». È un dovere che tutti dobbiamo sentire come un assillo. Con disciplina ed onore, dando il meglio di sé in ogni circostanza, per l'obiettivo più importante per il quale ogni donna o uomo delle istituzioni, come tutti noi membri del Parlamento siamo, possa lavorare. Tutelare la vita e la salute delle persone il nostro bene più prezioso. Io sono certo che insieme ce la faremo.

le informative, la rendono simpatico ai miei occhi, ma credo anche agli occhi di molti altri cittadini. La lascerei impegnato un attimo con il collega Marcucci in questo momento, perché credo che sia più importante quello che avete da dirvi. Io aspetto.

vede in lei anche l'uomo solo al comando, che manda lei, perché è uomo pacato e quindi con lei i toni è difficile alzarli (e io glielo riconosco) per evitare di venire lui perché è lui il vero responsabile, è lui che dovrebbe essere lì, è lui che oggi ha generato tutto questo problema. Il problema dell'Italia, in questo momento, si chiama professor avvocato Conte, su questo non ci sono dubbi. Signor Ministro, ci sono meravigliose forme d'arte che fanno dell'improvvisazione la loro spina dorsale, il loro manifestarsi. Mi vengono in mente il jazz, il teatro e lo sport. Queste meravigliose forme d'arte si fanno carico dell'improvvisazione ed è bellissimo in realtà. Ci sono altri ambiti della vita in cui invece l'improvvisazione, secondo me, è un problema e dunque la questione è diametralmente opposta: per esempio la politica, e soprattutto la politica di Governo. Quando la politica di Governo, invece di avere come stella polare la pianificazione, la progettazione e la visione, si dà all'improvvisazione è un grosso problema e se nel primo caso, in qualche modo, si genera nel pubblico che assiste un sentimento di gioia e di soddisfazione, nel secondo caso non ci sono dubbi che vengano generati altri due effetti che sono la povertà e la disperazione. Il combinato disposto, signor Ministro...

ha generato, nell'ambito di cui mi occupo da vicepresidente di Commissione (quindi turismo, commercio, piccola industria e quant'altro), forse il peggiore dei drammi, anche perché le attività produttive, molte delle quali non hanno neanche potuto aprire - *tour operator*, agenzie di viaggio e mi viene in mente tutto il mondo della montagna che oggi credo abbia stimato in 30 miliardi

quando va bene, perché a volte è il 3, il 5, il 7 o l'8. Dunque le chiedo, Ministro, ma davvero crede, semplificando, che se fosse 100 euro il fatturato di un anno, con 5, 6 o 7 euro si possano pagare le bollette, l'affitto, i dipendenti e quant'altro e soprattutto ci si possa vivere? *(Applausi)*. Io credo di no, Ministro, ma credo che lo sappia perfettamente anche lei, anche perché in questa situazione si corre un grande rischio, cioè che anche Golia,

nel modo più assoluto. In quel caso che cosa succede? Il popolo, quando è toccato nel vivo, quando è affamato, protesta. Mi rivolgo anche alla parte opposta alla mia: il popolo protesta e si sa bene cosa vuol dire protestare. Quando gli si impedisce di protestare nelle piazze, a volte magari usa i forconi

che possono avere le risorse e la possibilità di mettere in condizione tutti di poter essere serviti in sicurezza. È drammatica questa cosa.

Gli abbiamo anche fatto produrre le mascherine, gliele abbiamo comprate, abbiamo detto alle nostre aziende di riconvertirsi perché avevamo bisogno di mascherine, e poi le abbiamo comprate dai cinesi, ma questa è tutta farina del vostro sacco. sacco. Penso anche alla preoccupazione delle Forze dell'ordine perché quei denari lì molto probabilmente sappiamo da dove arrivano, sappiamo cosa sono, capiamo perfettamente se sono trasparenti? Qual è il problema dell'inquinamento di questi capitali? Non lo so. Sono risposte che non avete e non le avrete mai probabilmente, come non le avete mai avute per le nostre attività produttive. Signor Ministro, è veramente triste dirlo - e mi avvio a concludere - ma voi siete uno sciagurato Governo che ha generato solo tre cose: improvvisazione, povertà e disperazione. Concludo con una citazione dell'ex onorevole Mastella: tranquilli, bimbi, i responsabili...

Signor Presidente, colleghi, Ministro, l'approccio che il Governo continua ad avere nella gestione pandemica è sempre lo stesso. È trascorso quasi un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, ci si appresta a una nuova proroga, gli esperti ci informano che, fino a che non avremo vaccino in abbondanza, le fasi dell'epidemia continueranno a succedersi, ma la situazione rimane la stessa: venite a comunicarci il contenuto di decisioni già prese *(Applausi)*, che naturalmente sono già nelle mani dei giornali, con le veline di Casalino, e facendo finta di aspettare che il Parlamento vi dia le indicazioni per le decisioni finali. Ministro, la ringrazio della sua attenzione. Molti di noi si sono chiesti cosa avrebbero fatto al suo posto; sinceramente pochi sarebbero riusciti a gestire la prima fase dell'epidemia, considerata la prepotenza del virus; ma è trascorso un anno, e in questo anno, soprattutto noi di Forza Italia, in molte occasioni, non le abbiamo mai fatto mancare supporto e idee. Il presidente Berlusconi per primo le ha più volte espresso la nostra solidarietà per le decisioni che stava prendendo; ma, come ben sa, la pazienza ha un limite, e da lei ci saremmo aspettati almeno le scuse per aver presentato solo ieri *(Applausi)* la bozza del piano pandemico, che i suoi consulenti le avevano evidentemente nascosto nelle stanze segrete; piano pandemico che chiediamo da mesi, e solo grazie alle inchieste della magistratura e dei giornalisti scopriamo che in realtà era un copia e incolla di vecchie versioni. Andrebbe concessa un'onorificenza a Zambon, il ricercatore che non si è piegato alle minacce, e certe persone non dovrebbero più sedere ai tavoli decisionali che riguardano la sicurezza e la salute degli e le dirò che proprio tra i suoi alleati di Governo, i 5 Stelle, in 40 hanno chiesto la rimozione del segretario generale Ruocco. Abbiamo letto le notizie di stampa, valuteremo la bozza del nuovo piano pandemico. Ministro, lei poco fa ha invitato all'unità: certamente, in un momento così drammatico è fondamentale, ma invocare l'unità non significa nascondere le proprie responsabilità. È dal 2006 che il piano pandemico non viene aggiornato, quindi la colpa non è tutta sua, ma ormai avrebbe anche dovuto vigilare e far venir fuori la verità anziché infastidirsi con chi gliel'ha chiesto. Le diamo atto che un nuovo testo adesso c'è, anche se è una bozza con contenuti discordanti: ad esempio, leggendo un articolo del «Corriere della Sera» di si vede nel copia e incolla che il Ministero dovrebbe avere le dosi di farmaci antivirali e sono quelle 40 milioni di dosi che aveva ordinato il ministro Fazio nel 2011, ma magari è una piccola svista. Capisce bene che esiste una sola parola: vergogna. Ha fatto discutere l'inserimento di un capitolo sugli aspetti morali: faremo scegliere chi curare o meno? Leggo testualmente: i principi di etica possono consentire di allocare risorse in modo da fornire trattamenti non necessari a quei pazienti che hanno maggiori possibilità di trarne beneficio. È questo quello che lei ha appena affermato dicendo che non dobbiamo lasciare andare i più deboli? Non lasciamo indietro i più deboli e sul piano pandemico c'è scritto che curiamo solo chi può trarne beneficio? Voglio pensare che allocare risorse si riferisca a risorse umane (medici e infermieri) e non economiche, perché allora siete veramente indegni, se non usate il MES sanitario,

di questo tipo darà adito a tanti di quei contenziosi che nessuno prenderà più una decisione? E, se questa è l'intenzione, le centinaia di decreti legislativi che servono per dare attuazione alle leggi - 180 sono solo quelli riferiti a questa emergenza, 180 decreti attuativi che mancano per poter applicare le leggi già pubblicate

lavorano lì da anni, mentre nel nuovo bilancio è prevista praticamente l'assunzione di altri dirigenti, per cui in Agenas non si sa bene chi, cosa e come farà, ma in compenso ci sarà un dirigente ogni sei dipendenti. Complimenti, direi. Venendo al futuro prossimo - che poco roseo ci sembra, considerato lo stato della maggioranza, sempre che ci sia ancora - la ringraziamo per l'annuncio di 18 miliardi del *recovery fund* per la sanità, se erano già presenti nella vecchia bozza, visto che la parte riferita all'edilizia sanitaria rientrava in un capitolo diverso e non compariva quindi negli interventi specifici. Ottimo lavoro. Il gioco delle tre carte ha funzionato peccato che lei abbia ammesso che per la sanità di miliardi ne servano 60 e non sappiamo in che modo arriveranno, a meno che non abbiate deciso di utilizzare finalmente i soldi del MES sanitario, dopo aver fatto digerire i nuovi ingressi nella compagine ministeriale. confusione sulle zone (gialle, arancioni, rosse, bianche) e confusione sulle dosi di vaccini a disposizione, nonché sul controllo di chi riceve i vaccini. Ad esempio, chi monitorerà le vaccinazioni? L'Aifa, la farmacovigilanza? È dal 2017 che aspettiamo che ci sia un'anagrafe vaccinale in tutte le Regioni italiane.

sono arrivate tardi ed erano sbagliate, come ha appreso dai telegiornali tutta l'Italia. Che fine hanno fatto poi i 2 milioni stanziati per il personale del «112» impiegato nell'attività di contrasto all'emergenza i 50 milioni del cura Italia per gli interventi regionali finalizzati alla creazione di aree sanitarie all'esterno delle strutture ospedaliere? Molti pazienti, quelli fragili, che lei ricorda spesso, sono rimasti senza supporto. Sul tracciamento dei contagi non sappiamo niente. Noi chiediamo l'unità a tutti: ai pazienti che sono lasciati indietro, al tracciamento, alla *app* Immuni, ai ristoratori e ai baristi che aprono a giorni alterni e non sanno mai neanche cosa devono comprare: se il latte o niente. Fate presto, ha ribadito il presidente Berlusconi, ma usando la testa e provando a immedesimarvi in una delle famiglie che ha perso tutto. Ma voi, qualche volta, dai vostri Palazzi uscite? *(Il microfono automaticamente).* Signor Ministro, cerchiamo di avere meno *caos*. Aspettare è doloroso, dimenticarlo è peggio. Datevi una mossa. Se ci siete ancora, battete un colpo.

e uno su tre che la propria preparazione scolastica sia peggiorata. Nel 35 per cento dei casi, devono recuperare più materie dell'anno scorso. Ministro, c'è il problema concreto della dispersione scolastica. Il 28 per cento sostiene che, dall'inizio della pandemia, almeno un compagno nella propria classe ha smesso di frequentare la scuola. La stima è che almeno 34.000 studenti delle superiori a causa delle assenze prolungate potrebbero trovarsi a rischio di abbandono scolastico. Tutto questo, signor Ministro, non è confortante. Anzi, a preoccuparsene per primi sono proprio i ragazzi, che si sentono esclusi dalle scelte per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Il 65 per cento, addirittura, è convinto di pagare in prima persona l'incapacità degli adulti di gestire la pandemia. Il 43 per cento si sente accusato dagli adulti di essere tra i principali diffusori del contagio, mentre il 42 per cento ritiene ingiusto che gli adulti possano andare a lavorare quando a loro non è permesso di andare a scuola. Ministro, bisogna fare presto e attuare quegli interventi necessari per rendere la scuola un luogo in cui gli studenti possono svolgere l'attività scolastica in sicurezza. Quali siano questi interventi, signor Ministro, glielo dicono i ragazzi stessi. Sono loro che affermano che bisogna affrontare i problemi strutturali che affliggono da tempo la scuola. Pensiamo agli edifici scolastici, che non hanno spazi sufficienti e adeguati. Su questo tema, la Lega da mesi insiste per l'utilizzo degli spazi che le scuole paritarie potrebbero mettere a disposizione, oltre agli spazi di centri congressi, fiere, cinema e teatri. Pensiamo ancora alla carenza di organico rispetto al personale, altro tema sul quale la Lega da tempo si sta spendendo. Pensiamo al sistema di trasporto pubblico e alla mancata organizzazione per tempo di un trasporto dedicato agli studenti attraverso convenzioni con i privati. Ma non c'è solo questo, signor Ministro. In questa fase di emergenza sanitaria è fondamentale anche potenziare gli strumenti di prevenzione del contagio nelle scuole, a partire dai dispositivi di protezione fino al tracciamento. Mi permetto, signor Ministro, di sottolineare che ci sono anche impianti di depurazione dell'aria che potrebbero essere impiantati in molte nostre scuole.

è ciò che chiedono gli studenti e sono le stesse cose che da tempo chiediamo anche noi della Lega. Gli studenti hanno bisogno di certezze; questa situazione sta gravando sulle loro spalle, le diseguaglianze aumentano sempre di più e l'abbandono scolastico è un problema sempre più rilevante. Non possiamo lasciare nessuno indietro, soprattutto in un momento di crisi come questo. L'obiettivo di tutti e di tutte deve essere quello di riaprire la scuola in condizioni di totale sicurezza e in modo che sia accessibile a tutti gli studenti e le studentesse. Tutto questo, signor Ministro, si chiama programmazione, una variabile sconosciuta a questo Governo che continua a mettere toppe, a inseguire i problemi e a non aggredire, anticipare, prevenire; una parola, questa, che vi piace molto, ma che non sapete applicare nella realtà. Ministro, deve ammettere che quest'estate si è perso tempo e possiamo anche dare la colpa al comportamento irresponsabile degli italiani. Ma il comportamento maggiormente irresponsabile è stato il vostro, che avete preferito pensare ai banchi a rotelle e ai monopattini piuttosto che mettere all'opera aziende e operai per adeguare la scuola, dando in questo modo anche lavoro. Mi consenta inoltre, signor Ministro, di parlare della cultura e di tutto quello che si sta perdendo in questi mesi con musei, mostre, cinema e teatri chiusi. Le ricordo che con la legge di bilancio sono stati accolti ordini del giorno sottoscritti dal Gruppo Lega per la riapertura dei musei; mi auguro che anche per questo, per quello che lei ha detto oggi, possa essere mantenuta la promessa. Apriteli! Non penso che all'interno di musei e mostre si possano creare *movida* e assembramenti, che nei musei non ci sono mai stati. Apriteli! Date respiro alla nostra cultura, che sta per morire come stanno morendo le compagnie teatrali. Abbiate almeno la decenza di finanziare spettacoli in *streaming* e non di favorire Netflix. Questo è necessario, prima che tutti si dileguino *(Applausi)* e che non resti niente di un capitale culturale e umano che, se non viene opportunamente...

onorevoli colleghi, il virus continua a correre veloce; la comparsa di nuove varianti con maggiore capacità diffusiva, anche se con invariata azione patogena, ha semplicemente accelerato questo processo. Lo constatiamo semplicemente anche osservando quanto accade negli altri Paesi europei, che infatti alternano provvedimenti e fasi meno restrittive con altre che si spingono fino a *lockdown* totali. Il nostro Paese, che vive inoltre anche le difficoltà della regionalizzazione del Sistema sanitario nazionale per effetto delle norme del Titolo V della Costituzione, nel difficile cammino della lotta al coronavirus, pur tra le enormi difficoltà contingenti, ha cercato di mantenere sempre il giusto equilibrio tra restrizioni e concessioni, tra aperture e chiusure, pur considerando le grosse problematiche e le tante ripercussioni che ogni provvedimento portava con sé. Non dobbiamo mai dimenticare, però, un punto fondamentale e che tanti cittadini richiedono: la tutela della salute viene prima di ogni cosa. La salvaguardia dell'integrità e della vita di ognuno va oltre quelle che possono essere le richieste, anche giuste e motivate, di alcuni. Nessuno ha mai dimenticato, nei vari provvedimenti adottati, le conseguenze economiche, sociali e le complesse problematiche per tanti cittadini che essi avrebbero provocato, cercando di dare però sempre risposte concrete. La volontà politica è stata sempre quella di tutelare le fasce economiche più in difficoltà e i soggetti più fragili e vulnerabili del nostro stato sociale. Purtroppo, ad una maggiore elasticità e ad una riduzione delle misure più restrittive corrisponde, quasi come una logica conseguenza, un rapido aumento dei contagi, un'accelerazione della diffusione del virus e una sua impennata con la risalita dell'indice RT. Proprio in quest'ultimo periodo abbiamo avuto la dimostrazione di tutto ciò, la risalita e il raddoppio dell'indice di contagiosità dopo il periodo natalizio, che sicuramente è stata conseguenziale agli assembramenti e agli atteggiamenti superficiali e poco consoni alle raccomandazioni ricevute. Sempre di più occorre insistere nella continua sensibilizzazione ed informazione dei cittadini, nel richiamo al loro senso civico e di appartenenza alla collettività. Se non riusciamo a fare tutti questo processo di maturazione e di elaborazione interiore, non riusciremo a debellare o sconfiggere il virus. Qualsiasi provvedimento, anche il più condiviso e partecipato, necessita dell'adesione convinta di ogni cittadino. Si tratta di un'adesione che per la maggior parte c'è stata e di cui non possiamo che ringraziare gli italiani. È fondamentale ricordare che le norme si applicano e si realizzano completamente solo se ciascuno di noi comprende che, in questa pandemia, ognuno deve fare la propria parte ogni giorno, non per il semplice obbligo o per il timore di sanzioni, ma perché i nostri comportamenti responsabili sono una condizione indispensabile nella difficile battaglia contro il coronavirus. Chi governa deve saper centellinare e bilanciare le misure con i giusti equilibri. Se il virus è così dinamico e mutevole nella sua aggressività, anche le scelte politiche conseguenziali non possono essere statiche, ma devono essere equilibrate e modificate in rapporto all'andamento della pandemia.

che prevede misure meno restrittive rispetto all'area cosiddetta gialla, sempre al fine di assicurare la massima coerenza tra lo scenario epidemiologico riferibile a ciascun territorio e il grado di rigore delle misure di contenimento ivi applicato. Questa novità, concordata con il comitato tecnico-scientifico, rappresenta e racchiude, in questo momento particolare, più che altro un valore simbolico e un messaggio di incoraggiamento agli italiani: essere più virtuosi e attenti si può e si deve. Il secondo aspetto riguarda l'abbassamento del valore soglia degli indici di contagio RT, per entrare o passare nelle varie zone. Si tratta di un accorgimento di prevenzione, resosi necessario per arrivare prima del virus, con misure più restrittive, capaci di prevenire situazioni più difficili e critiche. Sicuramente un supporto fondamentale nella gestione di questa pandemia è iniziato con la somministrazione dei vaccini, la cui disponibilità progressiva ci permetterà di avere un'arma letale nei confronti del virus, a cominciare da chi è in prima linea, come il personale sanitario, e dai soggetti più deboli e fragili della popolazione. Le decine di migliaia di morti, le sofferenze delle terapie intensive, gli sguardi persi nel vuoto di chi sa che forse non ce la farà costituiscono un monito per istituzioni e cittadini, a cercare di fare sempre di più e meglio, nell'interesse della collettività. I tanti sacrifici richiesti, a cui tantissimi hanno aderito, con consapevolezza e coscienza, non possono essere vanificati nel momento in cui, pur tra i tanti dubbi e le tante incertezze, con la campagna vaccinale appena iniziata

Il Governo non nasconde la delicatezza della situazione sanitaria ed economica e si dice preoccupato che nel Paese possa avanzare da un lato un ingiustificato sentimento di scampato pericolo e dall'altro il rifiuto di nuove misure tese a contenere il numero dei contagi e, più in generale, la circolazione del virus nelle sue diverse varianti, autoctone e importate. Se questo è vero, non dobbiamo però nasconderci che ad oggi mancano un'esatta misurazione, un bilancio affidabile, un resoconto univoco e inattaccabile di quanto è accaduto sui vari fronti della crisi nel corso dell'ultimo anno. Lo sforzo al quale dobbiamo tendere - Parlamento, Governo, Regioni, sistema degli enti locali - è quello di attivare banche dati certificate e trasparenti, attraverso le quali l'opinione pubblica possa seguire l'evoluzione della pandemia, le misure e gli effetti delle stesse che gli organi decisionali hanno via via assunto, assumono e assumeranno. È dunque urgente un'operazione trasparenza sulle misure di prevenzione quali quelle enumerate dalla nuova azione che il Governo si appresta a perfezionare e su quelle legate all'assistenza sanitaria e alla campagna vaccinale in atto. L'autorizzazione del vaccino di Moderna, che si affianca quello della Pfizer, è una buona notizia ma non basta: serve una pluralità di soggetti affinché la campagna sia più celere, sistematica, equa e - appunto - trasparente. Dobbiamo comunicare con chiarezza che il vaccino è lo strumento per uscire da questo incubo collettivo che condiziona le vite di tutti, le relazioni, le dinamiche sociali, lavorative e affettive, che condiziona il percorso educativo e scolastico di un'intera generazione e per affrontarlo serve fiducia. Per generare fiducia serve trasparenza sulle responsabilità e sulla catena decisionale, sulla scelta delle priorità da dare, sulla sicurezza, su quali vaccini scegliamo di somministrare e perché, sul modello organizzativo, sugli esiti, sulla dimensione universale della vaccinazione per tutti e gratuita. Abbiamo cioè necessità di dare una prospettiva al Paese, di mettere una scadenza alla fase difensiva ormai in atto da un anno e proporre una visione attendibile di ripartenza in sicurezza. È infatti l'assenza di questa prospettiva, che pare ancora inafferrabile, a dividere in due il Paese tra chi è garantito e chi no, tra chi ha un reddito certo e chi se lo vede negare dalle restrizioni, tra chi riesce a esercitare il suo diritto allo studio e chi no. È l'assenza di prospettiva a rendere, al di là della buona volontà e dell'impegno dell'ottimo ministro Speranza e dell'intero Esecutivo, talvolta inefficaci i provvedimenti. È difficile, infatti, che chi non li condivide o se ne sente escluso, chi si sente ancora una volta trascurato li applichi di buon grado e se ne senta coinvolto.

a loro volta immediati, senza lungaggini burocratiche o intermediazione di soggetti economici terzi, che garantiscano ai soggetti interessati la sopravvivenza della loro attività economica e lavorativa e salvaguardino la loro dignità di cittadini e cittadine. Anche in questo campo possiamo e dobbiamo fare molto di più. Uno degli accenti che voglio porre non è però misurabile economicamente, anche se a volte alla condizione economica e lavorativa dei singoli è in qualche maniera collegato. Credo che il Governo tutto - e il Ministro della salute in particolare - debba farsi carico non solo dell'assistenza sanitaria e della salvaguardia economica, ma anche del benessere psicofisico dei cittadini e delle cittadine, in quest'anno fortemente messo a rischio dalle limitazioni che, giocoforza, abbiamo dovuto mettere in atto. Penso ai bambini e alle bambine, ai quali e alle quali il virus ha sottratto spazi e luoghi di svago e crescita; ai ragazzi e alle ragazze, la gran parte dei quali è ancora costretta alla didattica a distanza e di conseguenza, come pena accessoria, alla perdita di momenti di socialità, scambio di esperienze e crescita. alla didattica a distanza, apro una parentesi da uomo di scuola. Credo che questa sia un succedaneo che non potrà mai sostituire quella in presenza, legata ad aspetti che si aggiungono al mero scambio di informazioni tra docenti e alunni. La didattica a distanza va migliorata, pandemia o non pandemia, per integrare in futuro i nuovi modelli di didattica in presenza. Oggi siamo costretti a usarla in via esclusiva, spero ancora per poco. poco. Invece di dire che non funziona, mi aspetto che chi di dovere lavori per migliorarla quanto si può, valorizzando il grande impegno dei docenti che fanno spesso miracoli per reinventarsi una modalità

In questo senso - e chiudo la parentesi - apprezzo l'impegno enunciato ieri dal ministro Azzolina e sintetizzato dalla formula «ristori del sapere». Mi auguro che si tratti di un piano strutturato per integrare

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, è trascorso ormai un anno da quando il nostro *leader* Giorgia Meloni lanciò l'allarme sul rischio che veniva dalla Cina e il presidente Conte disse che non c'era da fare allarmismo, esponenti della maggioranza corsero ad affermare che bisognava abbracciare un cinese

Signor Ministro, oggi lei ci chiede e parla di unità e coesione. Ricordo che dalla parte politica di Fratelli d'Italia non sono mai mancate le proposte, che sono ferme negli atti parlamentari e nell'interpretazione di un ruolo politico che in questo ramo del Parlamento il

molto ricorrente in politica, ossia «lo avevamo detto», ma non credo che possiate essere convinti, oggi come ieri, di affermare che l'Italia sia stata un modello nel contrasto all'epidemia. Quest'estate pensavate che il Covid fosse un'esperienza archiviata e questo ha determinato un rilassamento che ci ha fatto piombare nella seconda ondata di contagi. Oggi, nella sua relazione, colgo elementi molto contrastanti: dice che vediamo la luce in fondo a questo tunnel, ma che è in agguato la possibilità di una terza ondata. Questo è stato l'atteggiamento oscillante privo di una strategia da parte del Governo che ci ha portato ad assecondare la corrente del contagio; e questo fallimento è diventato carne e sangue delle sofferenze degli italiani,

il mondo della cultura, per non parlare della scuola. Il ministro Azzolina per un anno ci ha detto che la Dad era la soluzione del problema; oggi ci dice che è molto preoccupata dalla mancanza di attività in presenza. Queste oscillazioni rendono l'esasperazione che il popolo italiano sta vivendo; e purtroppo, signor Ministro, non vediamo nelle sue parole nessun cambio di passo e nessuna assunzione di responsabilità rispetto al fallimento che si è già determinato. Il modello Italia non esisteva, lo dicono i dati, ora si aggiunge la vicenda dei vaccini, che pure era stata presentata come l'elemento risolutivo immediato, mentre oggi tutti capiscono che non è così.

che non ci sia un rapporto corretto: vengono usate come foglia di fico quando c'è da scaricare un fallimento, naturalmente quando si tratta di Regioni a guida amica,

in Campania, il cui governatore è l'unico politico e amministratore che si è autovaccinato.

di attivare i poteri ispettivi del Ministero, perché da due giorni un autorevole quotidiano, «il Quotidiano del Sud», parla letteralmente, con denunce circostanziate, di favoritismi nell'inoculazione dei vaccini a personale amministrativo che non è a contatto con il pubblico e a parenti di dirigenti sanitari. Quindi sì al vaccino, ma secondo le regole, come abbiamo detto tutti, dal Presidente della Repubblica in giù,

anzi, anche a questo proposito, che in Campania quegli eroi vengono trattati come profughi: ci sono foto del personale sanitario in fila sotto l'acqua e al freddo per essere vaccinati. Allora, non servono gli applausi e le testimonianze qui in Aula, quando nei fatti concreti la realtà che vive il Paese reale è ben diversa. Lei ha citato il grande Eduardo: «Adda passà 'a nuttata», ma molti cittadini pensano che più nera della mezzanotte non può essere.

oggi stiamo affrontando una materia importantissima e abbiamo ascoltato le comunicazioni del ministro Speranza, il quale ci ha detto percorso è ancora molto arduo e c'è una chiara ripresa della virulenza e della velocità di diffusione del virus. Ce lo dicono i dati del Regno Unito, della Germania, della Francia e addirittura della Svezia.

alle forze e alle risorse, per esempio, del volontariato, della Croce Rossa e delle tante associazioni di medici e infermieri volontari. Ho visto alcune esperienze a Milano che mi sono piaciute molto, perché lì il tampone costa troppo, quindi bisogna far sì anche che costi molto meno. Nel Lazio - dove siamo fortunati, sostanzialmente - e in Sicilia il prezzo è calmierato. Non dico di calmierarlo ma perlomeno di tenerlo basso, in modo tale che possa essere accessibile che quindi possa essere un'attuazione del diritto alla cura, di cui pure lei ha parlato, signor Ministro. Tale diritto alla cura è sancito dall'articolo 32 della Costituzione e vede correttamente anche la possibilità per i privati di fare profitto, ci mancherebbe altro.

bassi i prezzi dei tamponi. Si tratta di una misura necessaria per contenere e rallentare la velocità di diffusione del virus.

Allora - come ci dicono gli scienziati da mesi, da quando a giugno sono stati messi a punto i tamponi rapidi, che sono banali e sostanzialmente utilizzabili con banalissime competenze di carattere tecnico, più che scientifico scientifico - si diffondano e si trovino in ogni angolo della strada, delle nostre città e nelle varie piazze. Ci sono tantissimi volontari che avrebbero in mente l'intenzione di farlo però trovano ostacoli burocratici:

In questo senso, auspico che il ministro Speranza voglia esprimersi favorevolmente rispetto alla risoluzione che abbiamo presentato.

perché dall'inizio di questa terribile crisi non ha mai fatto mancare la sua presenza nelle Aule parlamentari per aggiornarci sull'andamento dell'epidemia e sulle decisioni conseguenti. *(Applausi)*. Ritengo sia una dimostrazione di grande responsabilità, della quale dovremmo essergli tutti grati. In tal senso, condivido ampiamente il suo invito all'unità e alla responsabilità: le due parole chiave che soprattutto oggi, grazie al vaccino, ci consentono di guardare con maggior fiducia al futuro. Ciononostante, questi sono giorni particolarmente difficili. Purtroppo, la pandemia - qui, come nel resto dell'Europa - è nuovamente in fase espansiva. Riteniamo dunque ampiamente condivisibile l'approccio

l'aggravarsi della pressione sulle strutture sanitarie. Per riuscirci, dobbiamo interrompere la trasmissione del virus, che può essere grave e pericoloso, soprattutto se contratto in forma aggressiva. Le centinaia di morti che si registrano nel doloroso e tragico bollettino quotidiano, a cui non dovremmo mai abituarci, sono lì a ricordarcelo costantemente. È dunque necessario, in ragione del peggioramento di tutti i parametri, prorogare lo stato di emergenza, al fine di confermare e rafforzare le misure di contenimento della diffusione. È una battaglia lunga, che sta mettendo a dura prova i cittadini. Per questo è auspicabile che, nell'ambito del modello dinamico per fasce, si favorisca una maggiore tempestività nell'accesso delle Regioni che presentano parametri particolari di rischio, ma contestualmente si introduca un livello di rischio inferiore a quelli fino ad ora contemplati. Precauzione e proporzionalità dovrebbero essere le parole a cui continuare ad ispirare la nostra azione. Purtroppo, la recrudescenza dei contagi potrebbe costringerci a prolungare o introdurre nuove limitazioni per le attività produttive. In tal senso, ci sembra necessario - e il Governo si sta già muovendo in questa direzione - approntare tutte le misure di ristoro necessarie per le categorie già duramente colpite da quasi un anno di inattività. Ministro, sa bene che questo virus ha acuito e allargato le disuguaglianze, colpendo con maggior ferocia le persone più fragili e in difficoltà. Nei prossimi mesi sarà necessario mettere in campo tutte le iniziative necessarie per ridurle, a partire dall'accesso al sistema sanitario.

molte persone non autosufficienti non hanno potuto avere accesso alle terapie; in particolare, quelle affette da disturbi mentali e fragilità psichica non hanno potuto essere seguite. Dunque, se rispetto a un anno fa abbiamo più medici, più infermieri e più posti in terapia intensiva abbiamo messo 12 miliardi aggiuntivi nella sanità, sappiamo che serviranno ulteriori investimenti. Penso soprattutto alle aree del Paese in maggiore difficoltà, quelle con un sistema sanitario nel quale i problemi esistevano già prima che arrivasse il Covid. Colmare questi divari e rimettere nel sistema le persone più fragili: questo dev'essere il nostro primo impegno.

La scienza e la ricerca hanno fatto straordinari passi in avanti, tuttavia - sono le sue parole - non abbiamo ancora vinto. Non dobbiamo dunque sbagliare la lettura di questa fase decisiva. Ora, infatti, arriva il momento più complesso, quello della somministrazione di massa: si tratta di un lavoro lungo e complesso, che coinvolgerà tutte le istituzioni e per il quale serviranno la massima collaborazione e una diffusa campagna di informazione. Il Paese è pronto ad aumentare il numero delle somministrazioni da effettuare, appena saranno autorizzati i nuovi vaccini. In tal senso e alla luce del mio accenno sulla necessità di tutelare le persone più fragili, le chiedo, signor Ministro, di formalizzare quanto prima l'impegno preso dal commissario Arcuri sulle vaccinazioni prioritarie alle persone con disabilità e ai loro *caregiver.* Sarebbe davvero importante chiarire definitivamente questo aspetto. Le persone con disabilità hanno sofferto più delle altre gli effetti del Covid e spesso sono state lasciate sole. Ora è necessario tutelarle, alla stregua di tutte le altre persone fragili. Mi avvio alla conclusione, dedicando qualche altro minuto una questione che mi sta particolarmente a cuore e che è indicata tra gli impegni che chiediamo al Governo: parlo della scuola. Ci voleva la pandemia - lo dico senza alcuno spirito polemico - per mettere la scuola al centro del dibattito pubblico? Questo forse sarà uno dei pochi aspetti positivi che la crisi sanitaria ci lascerà. Il nostro Paese, al pari di molti altri, ha dovuto fare i conti con una terribile incertezza, causata da una situazione del tutto inedita. In questi giorni, Nazioni come la Germania o la Gran Bretagna hanno ritenuto necessaria la sofferta decisione di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ogni Paese ha dovuto fare i conti con la difficoltà di tenere aperte le scuole in una situazione in cui la terza ondata non è più semplicemente un'ipotesi. Le scuole sono luoghi in cui, nonostante il grande lavoro di prevenzione fatto e l'impegno straordinario - che voglio sottolineare - dei dirigenti scolastici, del personale docente e non e degli studenti, ci si può contagiare. Dobbiamo continuare a lavorare in sinergia con le Regioni per consentire, alla luce dell'evoluzione del quadro epidemiologico da lei indicato con dati precisi, il ritorno in classe per il maggior numero di studenti. È del tutto evidente, infatti, come questa generazione stia pagando molto cara l'assenza di aule adeguate e, ancor di più, la mancanza di rapporti e relazioni. Serviranno ulteriori soluzioni, oltre al potenziamento dei trasporti e agli orari scaglionati. Ci dovrà essere per questa generazione un ristoro che possiamo chiamare cognitivo ed emotivo. Non sto parlando di un ristoro economico, ma di uno che è addirittura più importante. Occorrono quindi investimenti, iniziative, attività scolastiche di recupero, sostegni per ciò che è stato tolto a questa generazione in questi lunghi mesi, potenziamento dei servizi e delle reti territoriali, rinnovamento della didattica, come se quella a distanza potesse sopperire alla didattica in presenza, e quindi investimenti sui docenti e sulla loro formazione e servizi volti al benessere psicofisico. Solo per citare alcuni capitoli, serviranno risorse: il *recovery fund* ci darà la possibilità di disporne. Ora dobbiamo lavorare per preservare la capacità degli studenti di uscire da questa stagione con meno danni possibili, quindi mi auguro che si lavori per rafforzare gli strumenti che abbiamo, garantendo in via prioritaria il sostegno pedagogico e psicologico agli studenti, perché,

e, forse, soprattutto - uno quanto al disagio emotivo degli studenti smarriti, in cerca di senso per i loro giorni presenti e futuri, perché, se non riusciamo a costruire risposte, ci stiamo giocando il futuro dell'intero Paese.

ho chiesto di intervenire perché, francamente, avevo la necessità di rivolgerle direttamente alcune domande. Ho ascoltato tutte le sue informative nel corso

- e che bisogna stare a casa, perché c'è il problema della terza ondata. Questa è la verità. Signor Ministro, ha fatto un richiamo all'unità

quanto più possibile, sulla situazione e la seconda è la chiarezza, perché la maggior parte delle persone non capisce.

Piano piano, agli italiani è stato spiegato in modo abbastanza chiaro cosa significa (avrà visto che i dati sono cambiati).

per rimettere in piedi il sistema sanitario, affinché potesse affrontare la seconda e la terza ondata? Glielo chiedo perché, francamente,

il Governo abbia mai fatto una riflessione seria sul fatto che ci sono troppi virologi esperti che fanno una grandissima confusione nelle trasmissioni televisive, a cominciare da quelli che dovrebbero essere, invece, un supporto. Avete mai riflettuto sul fatto che forse una comunicazione univoca aiuterebbe tutti? Tanto, la medicina non è una scienza esatta. Spiegato questo alle persone, penso che possiamo anche cominciare a dare limiti alle uscite che generano confusione in una popolazione che, come sappiamo, è composita dal punto di vista della della cultura o comunque della capacità di apprendere questi temi. Penso sia doveroso. Ho ancora

che cerchiamo di richiamare l'attenzione del Governo su numerosi errori commessi rincorrendo la pandemia con la decretazione d'urgenza. siccome chi mi ha preceduto ha fatto un sunto più che significativo, vado oltre per aiutarvi a non fare altri errori. Non per voi, ma nell'interesse degli italiani. Mi riferisco principalmente al *vulnus* che si è creato non investendo in prevenzione sull'intera filiera e, soprattutto, in capitale umano debitamente formato, valorizzato e motivato. Personale medico e infermieristico che non solo talvolta viene sottopagato, ma reclutato addirittura in regime di somministrazione per attività routinarie come le vaccinazioni e talora remunerato con qualche credito formativo. modo, se da un lato si poteva parzialmente giustificare l'avere affrontato la pandemia come un nemico sconosciuto, perché evento raro e improbabile, quindi commettendo errori, dall'altro non è tollerabile che nella seconda e nell'ormai probabile terza ondata, generata da indecisioni e ritardi dovuti ad un albero decisionale che contiene nella sua linfa informazioni corrette, ma che usa in modo sbagliato, se ne possano commettere più che nella prima. Lo stanno a dimostrare gli oltre 570.000 attualmente positivi, l'aver portato i decessi a 80.000 e i posti letto di terapia intensiva occupati oltre la soglia critica. Così come un qualunque responsabile degli approvvigionamenti di una qualunque azienda sa dividere su sei possibili fornitori la commessa di un bene essenziale, ma non meno dovrebbe sapere che occorre privilegiare il fornitore che sia in grado di consegnare nei tempi più rapidi il prodotto con tutte le specifiche di efficacia e sicurezza richieste, anche a scapito della convenienza economica,

con i contratti ad oggi siglati possiamo vaccinare solo circa il 5 per cento della popolazione entro marzo e meno del 20 per cento entro giugno, in attesa delle 24 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca. Così come non aver diversificato le alternative nelle cure specifiche, a cominciare dai monoclonali disponibili e dal plasma superimmune con anticorpi neutralizzanti,

di terapie testate ed efficacemente utilizzabili sin dalla fine dell'ottobre scorso, solo che si fossero accettati i 10.000 trattamenti offerti da Eli Lilly per uso compassionevole, salvando potenzialmente almeno 10.000 persone: dunque, non solo vaccini. Ammesso che si continui a procedere in modo apprezzabilmente sostenuto, i primi risultati della profilassi vaccinale si avranno a primavera inoltrata e, siccome il Governo è sicuramente a conoscenza del fatto che l'emergenza economica genera vulnerabilità sociali e sanitarie non meno devastanti di quelle causate da un'infezione pandemica, avrebbe dovuto essere apprestata una strategia polistrumentale, dinamicamente aggiornata in ragione dei livelli di conoscenza acquisiti, in grado di aggredire il virus da tutti i punti di vista, anche dalla burocrazia dei cosiddetti decreti attuativi! Così come il ritardo maturato nella presentazione del piano pandemico speriamo sia colmato da tutte quelle indicazioni che ci aspettavamo da almeno sei mesi. Le misure di responsabilità individuale e collettiva, vale a dire l'uso delle mascherine, il distanziamento e l'igiene delle mani, in questa congiuntura avrebbero dovuto essere costantemente comunicate e divulgate con più efficacia, educando e sensibilizzando alla protezione per sé e per gli altri, sì da rendere del tutto ultronee prescrizioni normative che, invece, vi ostinate a perpetrare in modo ondivago, incerto e intermittente e che, con ulteriori cromatismi, può generare confusione.

senza continue proroghe dello stato di emergenza, capace di "convincere" per "non costringere". Purtroppo, ancora una volta, ci state dando prova del suo contrario.

il mito di Narciso è forse il più conosciuto della mitologia greca. Narciso era un giovane così tanto innamorato della propria immagine che perse la vita mentre si specchiava in un lago. L'invito che rivolgo a tutti noi in quest'Aula è quello di sapere andare al di là della nostra immagine, al di là delle nostre battaglie personali, e saper guardare tutti insieme al bene comune. Proprio stamattina, il nostro fondatore ha esortato tutte le forze politiche a stilare un patto trasversale con un obiettivo condiviso, riprendendo l'invito del presidente Sergio Mattarella a diventare costruttori di bene.

a dura prova da questo virus e da questa pandemia. Assistiamo ad un peggioramento generale dei dati epidemiologici. In queste settimane c'è un aumento dei contagi, un aumento dei ricoveri in terapia intensiva, un aumento dell'indice di trasmissibilità in tutte le Regioni. signor Ministro, noi, come lei, intravediamo finalmente la luce in fondo al tunnel. E intravediamo questa luce perché, in questi mesi, abbiamo avuto un faro importante, che è la scienza. La scienza, a differenza forse della politica, ha saputo lavorare con un obiettivo condiviso: i ricercatori di tutto il mondo hanno unito le forze per provare a trovare una cura oppure uno strumento di prevenzione contro questa infezione. un vaccino. Un vaccino che è stato prodotto con una tecnologia innovativa, una tecnologia mai utilizzata prima; un vaccino efficace per il 95 per cento, una efficacia altissima; un vaccino che, per la prima volta, sarà gratuito e disponibile per tutti coloro che vorranno vaccinarsi. Questo è un risultato straordinario, signor Ministro, così come straordinario è essere il primo Paese in Europa per numero di vaccinazioni somministrate. Abbiamo superato le 800.000 dosi di vaccino somministrato. In questa prima fase, come lei ha ricordato, stiamo vaccinando gli operatori sanitari, gli operatori e gli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), tutti gli ultraottantenni; poi partirà la seconda fase, in cui verranno vaccinati tutti gli operatori dei servizi essenziali, tutti i soggetti fragili; infine partirà la terza fase, quella della vaccinazione di massa, per la quale sono già previsti dei mezzi e degli strumenti straordinari. Adesso però dobbiamo continuare a credere nella scienza e nei dati che essa ci fornisce. Dobbiamo continuare ad investire nella scienza forse più di quanto è stato fatto finora, se pensiamo che l'Italia è il Paese col più basso numero di laureati ed è uno dei Paesi con il più basso numero di ricercatori: abbiamo solo quattro ricercatori per 1.000 abitanti, meno della metà della media europea. L'Italia è il Paese in cui il dottorato di ricerca, che è in assoluto il più alto titolo accademico, in alcuni concorsi non viene nemmeno valutato.

prevista per le zone con un basso numero di casi (meno di 50 casi per 100.000 abitanti, con un indice RT minore di 1). Questo barlume di speranza io lo colgo nella riapertura delle mostre e dei musei

cenno sulle scuole. I giovani sono coloro che hanno pagato a caro prezzo le conseguenze di questa pandemia: hanno dovuto rinunciare alla socialità, agli abbracci, ai primi amori; hanno dovuto rinunciare a vedere i nonni. Eppure, con grande spirito di responsabilità, hanno capito che il distanziamento era un atto di cura,

tra lo Stato centrale e le Regioni sia sempre più efficace. Troppe volte in questi mesi le disposizioni centrali non sono state attuate a livello regionale; in questa fase è quindi fondamentale la collaborazione a tutti i livelli istituzionali. Sempre sulla collaborazione si deve basare anche l'attuazione l'attuazione dei progetti previsti dal *recovery plan.* Noi siamo molto orgogliosi del piano che riguarda la sanità, perché i progetti su tale materia si basano su quelli che per noi sono i pilastri fondamentali: il rafforzamento della medicina territoriale, istituendo finalmente in tutte le Regioni le case della salute, gli ospedali di comunità, rafforzando la presa in carico domiciliare, fornendo ai medici di medicina generale gli strumenti di telemedicina che noi chiediamo da un anno (quanto sarebbero serviti già nella gestione di questa pandemia). Il secondo pilastro, per i progetti di sanità inclusi nel *recovery plan*, concerne le nuove tecnologie e la digitalizzazione: si parla da quindici anni di fascicolo sanitario elettronico, di cartella elettronica, adesso devono diventare realtà. investimenti in prevenzione: abbiamo detto in tutte le lingue che per passare dalla medicina d'attesa alla medicina d'iniziativa bisogna prevenire le malattie. Anche in questa pandemia i malati oncologici, i malati fragili sono spesso stati abbandonati perché non hanno avuto accesso a percorsi differenziali.

la storia non ci perdonerà se in questo momento non saremo in grado di costruire il nuovo Paese, il Paese che ci aspetta.

dai senatori Iori, Pirro, Errani, Garavini e Steger, n. 3, dai senatori Richetti e Bonino, e n. 4, dai senatori Bernini, Romeo e Ciriani. I testi sono in distribuzione. Ha facoltà di intervenire il ministro della salute, onorevole Speranza, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, sui vaccini l'Italia è partita bene, ma come il ministro Speranza ha ricordato, questa è una maratona che si vince rendendo perfetta non solo la macchina degli approvvigionamenti, anche quella delle somministrazioni. Su questo ha ragione chi popone strutture aperte ventiquattro ore su ventiquattro, perché non bisogna perdere un solo minuto e una sola possibilità di somministrazione. La sensazione è che, da quando è partita la campagna vaccinale, molti dubbiosi abbiano cambiato idea e che quello scetticismo che aleggiava in alcuni piccoli segmenti dell'opinione pubblica stia scomparendo. Per questo bisogna continuare con l'approccio da lei indicato, quello dell'ascolto e del confronto, evitando scontri tra tifoserie, che avrebbero conseguenze negative da tutti i punti di vista. Aspettiamo fiduciosi medicines agency (EMA) autorizzerà il vaccino AstraZeneca, quel giorno vedremo davvero la luce in fondo al tunnel e pare, come ha detto il signor Ministro, che sia imminente anche la richiesta di autorizzazione da parte di Johnson & Johnson per il proprio vaccino, che ha il grande vantaggio di richiedere una sola somministrazione per garantire una protezione piena. Nel frattempo, però, bisogna continuare a gestire la situazione in maniera responsabile e con quell'approccio prudenziale, che da sempre ha guidato le decisioni del Governo. Certo, ci sono stati momenti in cui i cittadini hanno faticato a comprendere alcune decisioni, soprattutto quando all'ultimo momento sono state cambiate le carte in tavola, quando non c'è stata linearità nelle comunicazioni o quando alcune misure non sembravano rispondere a un criterio di proporzionalità. Nonostante ciò, crediamo che nel suo complesso il modello delle differenziazioni regionali abbia funzionato e che soprattutto sia adeguato per affrontare la fase che ci attende, una fase, cioè, in cui i contagi non scendono, c'è l'incognita delle varianti del virus, c'è il rischio che sulla seconda ondata si innesti subito la terza, come sta accadendo in altri Paesi. Una nuova ondata metterebbe a repentaglio la campagna vaccinale e questo noi non ce lo possiamo assolutamente permettere. quindi, le nuove misure con la condizione che, se aumentano le restrizioni, devono anche essere rafforzati gli aiuti. Fino ad ora è stato fatto uno sforzo importante, ma purtroppo non basta. Sono passati dieci mesi dalle prime chiusure, si tratta di un tempo insostenibile per la maggior parte delle imprese e degli esercizi commerciali che oggi combattono la loro battaglia per la sopravvivenza. Quindi, subito lo scostamento di bilancio, subito quell'anno bianco fiscale per i lavoratori autonomi, subito indennizzi che tengano conto delle perdite di fatturato, subito lo stralcio delle cartelle fiscali per le piccole e medie imprese, che in questi mesi non hanno potuto lavorare o hanno potuto lavorare solo in maniera limitata. Allo stesso tempo, signor Ministro, l'esperienza di questi mesi ci suggerisce che alcune deroghe rispetto a specifici contesti o situazioni sono necessarie e non rappresentano in alcun modo un pericolo. Mi riferisco al modello seguito durante le vacanze natalizie e confermato anche in questi giorni, con la possibilità di spostamento tra piccoli Comuni. è particolarmente vero in territori di montagna, dove la chiusura degli impianti di risalita sta diventando anche un problema per il presidio e quindi per la sicurezza del territorio. Venga concessa ai gestori la possibilità di aprire gli impianti, che senza turismo e senza spostamenti tra le Regioni avrebbe come unico effetto quello di distribuire ancora meglio le persone che salgono in montagna per attività motorie e sport individuali e che oggi, con gli impianti chiusi, tendono a concentrarsi in alcune zone. Si tratta, cioè, di rendere ancora più sicure attività all'aria aperta, con persone distribuite nel raggio di centinaia di metri, tutto molto meno pericoloso di una spesa al centro commerciale o di un sabato pomeriggio per le strade dello *shopping* cittadino. Chi non capisce queste ovvietà ovvietà non conosce la montagna o è mosso da un pregiudizio che purtroppo sta danneggiando inutilmente i nostri territori. Facciamo invece tesoro di quanto abbiamo appreso in questi mesi e che verifichiamo quotidianamente nei nostri territori, favoriamo quei comportamenti individuali e collettivi che non costituiscono un rischio e che rendono meno faticosa la vita delle persone e soprattutto accompagniamo queste nuove misure con un impegno senza precedenti per l'economia e per la campagna di vaccinazioni, che è la battaglia più importante, quella che ci guiderà fuori da questa drammatica esperienza. È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie alla risoluzione presentata dalla maggioranza. il Gruppo Italia Viva - Partito Socialista voterà sì alla risoluzione di maggioranza. Questo è il tempo della responsabilità di fronte alla pandemia, ma Ministro, che questa risoluzione sia davvero un punto di partenza per ricostruire la sanità e non navigare a vista come troppe volte il virus ci ha costretto a fare. La salute può e deve essere la forma più alta di democrazia e uguaglianza, senza nessuna differenza di età, genere, territorio, stato di salute e reddito. Questo ideale è quello che si configura nel Servizio sanitario nazionale che tante volte lei ha detto di voler difendere, giustamente. Ma troppe disuguaglianze e troppe falsità ancora circolano. Pensiamo alla scienza. Lei ha detto giustamente che la scienza è il nostro Quante falsità girano ancora sui vaccini, che non sarebbero sicuri perché il tempo a disposizione molto breve per arrivare a un vaccino avrebbe fatto saltare le fasi?

una medicina integrata a domicilio soprattutto per gli anziani. Il miliardo del *Recovery fund* per tre anni per fare genericamente una medicina integrata domiciliare è molto scarso rispetto alle esigenze. Io spero sempre che il Parlamento possa parlare anche di risorse

Inoltre, non è possibile che in una situazione di pandemia ci siano ancora dei precari nell'Agenas, tra i medici, il personale sanitario gli assistenti sociali. Guardiamo a questa pandemia come una grandissima opportunità per avere zero precari nei servizi sanitari e sociali. Personalmente ho proposto la costituzione di una guardia sanitaria nazionale in quanto abbiamo bisogno di prepararci a eventuali altre pandemie. Abbiamo pertanto bisogno di flessibilità (e non solo di costruzione di

di abbandonare altri malati; quindi dobbiamo assolutamente agire in questo senso. Signor Ministro, colleghi, noi dobbiamo riprendere la bellezza del quotidiano, perché le nostre vite sono stravolte. Per chi crede, il Papa domenica ha fatto un bellissimo discorso sul senso del battesimo di Gesù. Gesù è venuto tra noi per essere prossimo e riprendere il quotidiano. Lei ha fatto un appello all'unità e io rivolgo un appello a lei: per riprendere la quotidianità, la bellezza del quotidiano dei nostri concittadini, dobbiamo dare

sono andato a fare un po' di ricerche per parola chiave. La prima parola che ho immesso è "Arcuri". viene fuori tanta roba, signor Ministro. Viene fuori la vicenda delle mascherine e delle provvigioni pagate a persone di dubbia, conosciuta problematicità (provvigioni pesanti, evidentemente). Viene fuori la vicenda delle mascherine prodotte da FCA e risultate poi non conformi. Ministro, rispetto ai suoi ringraziamenti rivolti ad Arcuri e rispetto alla mia povera ricerca per parola chiave, viene fuori la vicenda dei ventilatori, ai quali la trasmissione "Report" ha dedicato un'intera puntata;

in un mese; Arcuri non sa che in Italia si producono circa 200.000 banchi all'anno. Continuando la ricerca su "Arcuri", signor Ministro, è venuta fuori la vicenda dei vaccini e delle siringhe

C'è da capire se è vero o non è vero che mister Arcuri deve restituire un milione e mezzo allo Stato, perché avrebbe ricevuto un milione e mezzo in più di compensi rispetto ai limiti di legge. Ministro, mi perdoni, ma il suo ringraziamento è una goccia nel mare rispetto a quanto lo Stato ringrazia il supercommissario Arcuri e,

Dopo è venuta fuori la vicenda dell'unità che cercate sulle azioni e sul fatto che bisogna fare i vaccini. Benissimo, Ministro, credo che nessuno dei parlamentari dell'opposizione si spertichi o si arrampichi sulla circostanza che non bisogna vaccinarsi. Semmai, cercate negli altri banchi, dove siedono ancora i nostalgici di quei bei movimenti no vax e no tutto. Cercate di là

rispetto a quanto sta accadendo nel Paese, le posso affermare adesso, senza timore di smentita, che questo non è un Paese unito; è un Paese martoriato, diviso e prostrato

Dovete essere orgogliosi del *record* di abbattimento di PIL rispetto a tutti gli altri Paesi europei? Ministro, per questo c'è da chiedere solo scusa e, infatti, Google, che è bravissimo, riporta due pagine. pagine. Ministro, questi due parametri che le ho dato (*record* di decessi e *record* di abbattimento di PIL) in realtà sono il voto dell'esamino

infatti, alle misure di contenimento, restrizione e privazione delle libertà di impresa e individuali. Ministro,

non sono stati fatti i test. Lunedì scorso lei ha riferito che la settimana passata è stata caratterizzata da un grave peggioramento di tutti i parametri. Lunedì Lunedì scorso abbiamo fatto 90.000 tamponi; in Inghilterra fanno 500.000-600.000 tamponi al giorno

È un'azione talmente banale da fare, realizzandola su numeri consistenti, che non si capisce cosa state facendo con questa mappatura del virus. Non avete fatto Non avete fatto i protocolli per le cure domiciliari per i medici di medicina generale. Non tenete sotto controllo quello che sta facendo l'Aifa, che sembra la bella addormentata nel bosco. Non viene neanche in audizione in Commissione perché non ha tempo. Non avete fatto il piano pandemico, che ci avete consegnato l'altro ieri, sul quale avete scritto cose inenarrabili. Non avete fatto e regolato i trasporti per consentire di riaprire le scuole nel momento in cui è acclarato che la seconda ondata è stata causata proprio da tale problema. E allora, Ministro, sull'altro versante, quello che voi vi accingete ora a replicare, incrementare e

perché, dopo un anno di azioni di costrizione e di restrizione delle libertà individuali, queste misure non funzionano più e non funzioneranno più. Dovete mettere mano alle altre misure, quelle del contenimento sanitario. I due campi su cui voi avete meritato il voto, hanno come misura, due parametri. Quello del contenimento con le misure sanitarie

è giudicato dal *record* dell'abbattimento del PIL. Voi avete fatto il massimo sulla possibilità di costringere gli italiani a non esercitare le proprie libertà con un danno gigantesco sul PIL del Paese e il minimo rispetto alla protezione sanitaria dei nostri concittadini. In conclusione, Ministro, rispetto a tutto questo, le suggerisco che le suggerisco che non sono i numeri che io ho elencato, che da soli dicono e certificano il fallimento di quanto lei ha fatto; non è Renzi che vi manda a casa, come abbiamo ormai capito; non è neanche il Covid che vi manda a casa: sono gli italiani che non ne possono più e vi manderanno a casa appena gli sarà data la possibilità di farlo.

ma io sfido chiunque a dimostrare che in una vicenda così drammatica ci sono coloro che hanno le risposte già pronte.

provare a indicare i tre punti su cui dovremmo tutti riflettere. Il primo: i vaccini. È chiaro che con i vaccini si apre una condizione nuova, una prospettiva positiva. A tal proposito, i commenti dei primi giorni dell'avvio della campagna vaccinale si sono dimostrati non puntuali, per usare un eufemismo. Tutti i commenti dicevano che avevamo già fallito anche la campagna dei vaccini, ma i risultati per ora sono positivi. Lo dico aggiungendo che non bisogna fare - come giustamente il Ministro nella sua comunicazione non ha fatto - del trionfalismo.

l'immunità di gregge. Bisognerà prestare grande attenzione e avere una capacità organizzativa che dovrà impegnare tutti; bisognerà avere una capacità di convinzione. E poi - come giustamente è stato detto - certe funzioni pubbliche esigono coerenza: un operatore di una RSA decide di non vaccinarsi, è legittimo, ma deve scegliere di non operare più in fare della polemica ideologica, ma per un problema che - come abbiamo visto - è molto concreto. Su questo primo punto dobbiamo lavorare. Signor Ministro, penso sia giusto sostenere tutti gli sforzi di trasparenza sulla questione dei vaccini per consentire anche a chi non è

è indiscutibile. È inutile che continuiamo, a seconda delle posizioni, a chiedere aperture o chiusure È evidente che, se Paesi come la Gran Bretagna, la Germania e l'Olanda - praticamente l'Europa intera - stanno ulteriormente rendendo più una ragione ci sarà pure. Potremmo continuare a fare questa discussione senza soluzione di continuità. Possiamo dire che è responsabilità del Governo se i dati della pandemia sono in crescita? No:

per le vacanze di Natale, ero per una soluzione più rigida; capisco tutti i problemi, ma ero per una soluzione più rigida, questo è l'unico modo oggi di ridurre la crescita della pandemia. E non lo dico solo

a governare il processo di gestione della pandemia e, allo stesso tempo, affrontare la questione dei ristori.

e cioè sulla costruzione di un sistema di ristori fondato sul fatturato e sul meccanismo fiscale. Sapete che il Governo ha già detto che è disponibile a lavorare in questa direzione e potremmo dare certezze. Faccio questo ragionamento, rivolto in primo luogo all'opposizione, perché credo che elementi più critici siano la confusione e l'incertezza

sarebbe determinante per accelerare l'uscita dalla pandemia e, dunque, la ripresa e il rilancio economico.

ma di apertura di una fase nuova nel Paese. Su questo spero che si possa arrivare finalmente a non fare più gli stessi dibattiti. Lei, Ministro,

fare le vaccinazioni e a questo proposito apprezzo quanto detto dall'opposizione: nessuno è contro la vaccinazione. Deve uscire un messaggio di chiarezza. Da questo punto di vista, Ministro, personalmente penso che parlare di zone bianche sia un messaggio...

e ristori contro la crisi economica - potremmo provare a dare un messaggio positivo. Dopodiché la dialettica politica tra maggioranza e opposizione vada come deve andare.

cosa diciamo? Dobbiamo essere coerenti. Possiamo realizzare il passo in avanti? Lo spero e attendo sempre anche la minima apertura, perché per me ciò che importa davvero è dare certezza agli italiani, e non fare confusione. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

nostra; suggerimenti che ci pervengono ovviamente dal territorio, da tutti i cittadini che continuamente ascoltiamo in merito a tutto quello che sta succedendo. È passato un anno ormai da quando, per la prima volta, le autorità di Wuhan ci hanno detto - forse anche un po' tardivamente - che c'era un allarme di contagio rispetto a quello che, purtroppo, è diventato una pandemia globale che ci sta attanagliando ormai da troppo tempo. Abbiamo trascorso un anno pieno di sofferenze, paure, disagi sociali, economici e psicologici, ma la strada del ritorno alla normalità è ancora lunga: lo dicono gli scienziati, lo ribadiscono gli esperti. forse possiamo iniziare a intravedere una luce, perché abbiamo una speranza grazie agli sforzi portati avanti dalla ricerca scientifica, che finalmente ha illuminato la strada. Ma non abbiamo ancora vinto: il percorso non sarà breve. Devo ringraziare davvero, ancora una volta, in quest'Aula, tutti gli operatori sanitari che stanno salvaguardando le persone, che, purtroppo, sono colpite dalla pandemia. Il virus non ci sta lasciando neanche un momento e sta circolando ancora di più. Quindi, grazie davvero a tutti gli operatori.

deve essere reclutato. Signor Ministro, abbiamo sentito anche del suo nuovo accordo con i medici di medicina generale: benissimo, perché sono i nostri primi interlocutori, per cui, se anche loro hanno la possibilità

Il futuro è nel sentirsi fratelli e non nel voler dominare, ha detto Papa Francesco, e viene subito in mente l'immagine del Santo Padre in una piazza San Pietro vuota; immagine che si affianca a quella del nostro Presidente della Repubblica, quando ha detto che dobbiamo essere costruttori

Alla domanda specifica su che cosa abbiamo fatto di sbagliato, hanno risposto: quello che potevano fare le persone che non sapevano qual era la strada da percorrere. Quindi è stato fatto molto bene;

è stato fatto prima nell'emergenza, tutti noi ci abbiamo provato. Gli altri Paesi europei non stanno meglio di noi. Come sappiamo, siamo oggi tra le prime regioni in Europa per le vaccinazioni, per cui riusciamo ad affrontare anche questa emergenza.

e, solo limitando le cause dell'epidemia, saremo in grado di favorire anche la ripresa economica, e ne abbiamo veramente tanto bisogno. In tutto questo la somministrazione più veloce possibile del vaccino può consentire di tornare alla normalità in tempi brevi,

convinta che anche da questi segnali dobbiamo imparare. Bisogna essere pazienti e avere fiducia, tanta fiducia, anche e soprattutto nella scienza e investire soprattutto nella ricerca: è un altro messaggio che ci sta dando questa pandemia. Guardiamo che cosa siamo riusciti ad avere in poco tempo, grazie alla tecnologia innovativa dei vaccini

che ringrazio ulteriormente, debbano continuare a giocare un ruolo fondamentale in questa importante partita che è tutta della salute. *(Applausi)*.

e cerca anche, con uno stile che a noi piace, di affermare le proprie ragioni. Lei oggi ha fatto un intervento pieno di speranza, nel vero senso della parola, perché, in realtà, ha parlato prevalentemente del Piano nazionale vaccinale. Ha anche usato

ha affrontato, per quanto possibile "alla meno peggio", la situazione dell'emergenza sanitaria. Ha parlato più volte della necessità dell'unità nazionale e, quindi, dell'unità del Paese, affermando che solo uniti si può abbattere questo nemico invisibile, che la nottata non è passata, che

Sostanzialmente, poi, ella si è soffermato sul Piano nazionale vaccinale, affermando, tra l'altro - anche se poi ha detto che le graduatorie non le interessano - che, con 800.000 vaccini, siamo al primo posto 800.000 vaccini, siamo al primo posto in Europa. Io non so se veramente siamo al primo posto in Europa, ma penso che, purtroppo, andiamo ancora a rilento. Io

quello che per noi di Forza Italia appare giusto affermare oggi è che non è andato tutto bene. lo *slogan*: «Andrà tutto bene». Ecco, purtroppo, a distanza di circa un anno, siamo costretti ad affermare che non è andato tutto bene. La nostra è stata una opposizione seria e costruttiva, una opposizione di proposta e non di protesta. Anche se i due termini sembrano simili, in realtà sono molto differenti. Quello che noi affermiamo con estremo rammarico, tenuto conto dell'approccio che diamo alle problematiche del nostro Paese - a noi sta a cuore la sorte del popolo italiano è che in questi mesi, quando abbiamo avanzato proposte che poi sono risultate essere estremamente utili, purtroppo quasi mai sono state prese in considerazione, e talvolta sono state anche maldestramente respinte da una maggioranza che quasi sempre è stata sorda, perché ha ritenuto che tutto sommato era in grado di non sbagliare mai. E, invece, mi pare che così non è stato. A nostro giudizio, avreste dovuto chiedere scusa agli italiani in tante occasioni, perché tante sono state le cadute di stile.

la gestione di un percorso che si riflette su altre questioni: sulla scuola, sul trasporto pubblico locale, sulla vita delle famiglie. Questi sono temi che - a nostro giudizio - hanno

(il nostro esperto) - è soprattutto una questione di dati più che di date: non sappiamo esattamente quanti sono i contagi e i focolai nelle scuole; si parla soltanto di quando chiuderle o riaprirle. Esiste una possibilità di venire incontro a queste esigenze? Forza Italia ha fatto le sue proposte anche in questo caso; abbiamo proposto - per esempio - di fare in modo che possano essere riaperte stabilendo dei turni

Nella fase delle vaccinazioni bisognava pensare anche all'assistenza domiciliare e alla possibilità di effettuare i vaccini in casa *(Applausi)*, facendo in modo che tutto questo avvenga nel più breve tempo possibile, potenziando anche e soprattutto la medicina territoriale. Non è uno *slogan*: bisogna fare le cose. Degli anziani il signor Ministro si è fatto carico nel suo intervento, dicendo che sono la terza categoria che va sorretta e alla quale va rivolto il Piano nazionale di vaccinazione. Va benissimo, ma non dimentichiamo

Sappiamo che l'obiettivo è tenere la pressione ospedaliera bassa e ci sembra questa la strategia giusta da portare avanti. Signor Ministro - lo diciamo a tutta la maggioranza - per favore, scrivete regole chiare, ragionevoli e, soprattutto, comunicatele in modo tempestivo, perché la gente, oggi, con un giorno giallo, il giorno dopo arancione e il giorno fa confusione e non capisce più qual è la strada che deve seguire. *(Applausi)*. Questo è un grosso errore, perché nella confusione non riusciamo a far capire bene ai cittadini come bisogna muoversi e quali regole vanno seguite. Servono regole ragionevoli

all'ultimo momento, rischiate davvero di mettere ulteriormente in difficoltà delle attività che già sono al collasso. Comunicate prima le iniziative e le regole che volete portare avanti.

che si possano tenere comunque aperte delle attività magari con dei protocolli più stringenti: se un ristorante ha una metratura di 150 metri quadrati

anche nell'applicare le sanzioni nei confronti di coloro che non rispettano le regole. Sulla scuola, tutti hanno detto che è importante che i ragazzi tornino a scuola,

su misure quantomeno discutibili, ma programmiamo già adesso l'idea di riaprire le scuole fra un po' di tempo. Ministro, ascolti bene. Cinema, multisala, centri congressi e fiere sono spazi che possono essere utilizzati a sostegno della scuola. alle scuole paritarie, cerchiamo quella collaborazione tra pubblico e privato che consenta ai nostri ragazzi di avere gli spazi necessari.

Non entro nel merito degli aspetti organizzativi, perché non voglio fare polemica; l'ho detto fin dall'inizio, altrimenti sembra di tirare in ballo sempre le stesse situazioni. Ci sarebbero tanti argomenti, ma lasciamo perdere. strategia per ottenere una buona vaccinazione di massa. Lo so, Ministro, che lei è preoccupato, perché è un tema che non è stato trattato.

tutti a farci vedere che facciamo il vaccino. La corsa al vaccino crea insicurezza nella cittadinanza, in quanto qualcuno comincia a dubitare: come mai tutta questa corsa in tempi così rapidi, con vaccini che sono ancora

dando regole, portando rigorosità nel campo scientifico e magari organizzando delle trasmissioni televisive *ad hoc*.

è chiaro a tutti che in un mondo in macerie per una pandemia e una recessione che sembrano non aver fine, non c'è Governo in Europa in questo momento che non porti sulle spalle i crismi della impopolarità. Ministro Speranza, in questo momento non c'è alcuno che, al di là di quelli che possono essere gli interventi, voglia prendere il suo posto, in quanto ogni Governo deve assumere in questo momento delle decisioni terribili perché i tempi sono terribili. Gli amici inglesi, che hanno deciso di fare da sé, sono in recessione per la prima volta da undici anni: il PIL è crollato del 20,4 per cento nel trimestre aprile-giugno rispetto -

E non stanno meglio nemmeno i nostri amici francesi, che hanno dovuto registrare nell'ultimo periodo un crollo storico del PIL, il più grave dal Dopoguerra. Pensate che la contrazione che è stata registrata a Parigi ha raggiunto il valore *record* del 13,8 per cento, superiore a quella italiana. Per non dire poi della Germania, la tanto citata e decantata Germania, con Angela Merkel che è stata costretta qualche settimana fa a fare un discorso drammatico alla Nazione, con il peggior calo dell'indicatore del PIL dal 1970 e con un *lockdown* che nelle prossime ore forse diventerà ancora più severo e ancora più brutale per i cittadini tedeschi.

conti le pulci alle decisioni del Governo, magari cavalchi un po' anche l'onda delle tensioni sociali - vero senatore Ripamonti? - e continui a trattare i cittadini come fossero produttori di consenso elettorale. *(Applausi)*. Perché non iniziamo oggi davvero quella che tutti noi chiamiamo una svolta? Perché non decidiamo una volta per sempre di cominciare a ragionare diversamente e di cominciare a trattare i cittadini per quello che sono? persone da tutelare, persone da tutelare nelle loro famiglie *(Applausi)*, persone da tutelare nel loro posto di lavoro, persone da tutelare nella loro vita sociale, perché i dati

le persone muoiono, signore senatrici e signori senatori. Lo dico perché anche oggi ho sentito in questa Aula molte battute contro quel governatore, contro quel Ministro, contro quel sindaco, contro quel commissario. Ho sentito molti insulti e molte risate, ma fuori da questa Aula non c'è nessuno che ride. Non ridono le 2.636 persone ricoverate oggi in terapia intensiva, non ridono i familiari delle 3.492 persone decedute per Covid nell'ultima settimana; settimana; non ridono come state facendo voi. Da questa crisi dobbiamo capire che usciremo tutti più forti oppure tutti più deboli. Questa è una pandemia che non fa distinzione di colore politico e che non fa distinzione di rango, di censo o di latitudine; questa è una pandemia che ci lega tutti

ci sono milioni che non sono stati ancora spesi nei trasporti locali, nei tracciamenti, nelle USCA. Ma non importa; diamoci una mano, signori, perché dinanzi a noi il ministro Speranza vi dice che è in arrivo una terza ondata, che sta per travolgere il continente europeo. Questo vi ha detto oggi il Ministro; non è tempo dunque di dividerci, ma è tempo di collaborare, ciascuno con le proprie competenze.

dedicati alla sanità, anche grazie all'intervento e al contributo di Italia Viva, sono saliti a circa 20 miliardi, che si sommano ai 13 miliardi che questo Governo vi ha dedicato l'anno scorso. Stiamo parlando di risorse complessive per 33 miliardi, che è una cifra eccezionale per la sanità italiana. È eccezionale proprio perché nel decennio trascorso e precedente al 2018 la sanità ha avuto tagli per 37 miliardi, tradotti in ospedali chiusi e posti letto cancellati. I 33 miliardi complessivi dedicati alla sanità

qualsiasi tipo di richiamo a quei soldi che giacciono nelle casseforti di quell'organismo tecnico intergovernativo che non ha niente a che vedere con l'Europa e che si chiama MES. *(Applausi)*. Ci sono 33 miliardi e abbiamo fatto da noi. Non siamo andati nello Stato del Lussemburgo a chiederli; non ne abbiamo necessità.

Germania o la Francia, ma in proporzione alle capacità finanziarie della Francia e della Germania questo Governo ha messo in campo più soldi. Se l'Italia è ai vertici dell' Europa per numero di vaccini somministrati,

la parola «cittadini». Ci sono, però, in questo momento milioni e milioni di italiani che ci chiedono di concentrarci sulle cose reali che servono al Paese.

*blaming the victim* è un processo per cui una persona arriva a sentirsi colpevole. È una specie di autocolpevolizzazione. Nella crisi finanziaria, per esempio, le vittime dei *bankster* erano state colpevolizzate per avere vissuto al di sopra delle loro possibilità e sui giornali e nei *talk* era un trionfo di economisti che spiegavano che bisognava tirare la cinghia, che era arrivato il tempo dell'austerità come giusta espiazione. Con la crisi sanitaria si sta replicando lo stesso meccanismo di colpevolizzazione: è colpa dei cittadini che diffondono il virus, che si ammassano in centro, che bevono l'aperitivo, che addirittura vorrebbero il ritorno dei figli a scuola o che, addirittura, vorrebbero prendere i mezzi pubblici. Il virologo si sostituisce all'economista in una trama uguale. Insomma, è colpa delle persone che non si sono imposte l'auto *lockdown*. Il Governo fa quel che può; ci mette delle pezze colorate e ogni tanto dà la possibilità di uscire, ma solo per vedere l'effetto che fa e poterci poi dire: è stata tua la colpa, adesso che vuoi? lasciare la salute fuori dalla battaglia politica. No, ministro Speranza, lasciate la salute fuori dal *business;* il *business* delle mascherine - fa finta di non sentire - marchiate FCA o importate dalla Cina. Sono l'emblema della vostra sudditanza rispetto al potere. Ministro, lasciate la salute fuori dall'ingordigia delle multinazionali. Non è possibile che le multinazionali del farmaco scrivano contratti dei quali non si può sapere nulla nel dettaglio. I Governi pagano e buonanotte al secchio e in caso di danno da vaccino, Big Pharma è immunizzata da responsabilità perché gli avrete regalato sicuramente pure questa malleva totale. Il diritto alla salute non passa dal diritto di Big Pharma di ingrossare fatturati e profitti con i nostri soldi. Infine, ministro Speranza, non lasciate la salute all'incapacità e all'arroganza di Arcuri. Basta! Basta! Basta! Che penoso teatrino vedere questo Arcuri minacciare querele, tappare la bocca ai giornalisti con la schiena dritta, che vogliono solo sapere dello scandalo del traffico delle mascherine dalla Cina, dei costi gonfiati e di strane società di mediazione. Ancora una volta saranno i giudici a dirci chi si è fatto la «magnata» perché qui c'è odore di gran «magnata». Il Governo non sta onorando il diritto costituzionale alla salute degli italiani, anzi li sta infilando dentro il *blame victim* e così se qualche ristoratore o qualche negoziante vuole resistere all'inesorabile fallimento di impresa, al buio della disperazione... ...di colpe non sue, ecco che quel ristoratore deve sfidare le regole, i DPCM e la campagna mediatica. Speranza, un anno di vostra incapacità si riassume nella faccia di Arcuri, nelle mascherine di Elkann o dei cinesi, o nelle siringhe del prossimo che si farà i soldi grazie al Governo. Più che in emergenza, siamo alle grandi occasioni. Signor Presidente, fino all'ultimo non rinunciamo ad offrire agli italiani istituzioni che, anche in un momento non facile come questo, un modo di agire in Parlamento con modalità che secondo me sono profondamente sbagliate. Ho apprezzato molto, Ministro, il modo in cui lei oggi ha usato toni di gravità e serietà istituzionale. Se lo avesse fatto l'intero Governo in questi mesi difficili per tutti, ci saremmo evitati qualche guaio in più. Lei oggi ha fatto al Parlamento un appello alla responsabilità e all'unità. Mi permetta di accogliere il suo appello e mi permetta anche di rivolgere dall'opposizione al Governo un appello alla responsabilità e all'unità. Questo è infatti il momento nel quale il Paese non può vedere alcuna istituzione repubblicana agire con leggerezza e superficialità. Lo voglio dire perché siamo tutti consapevoli che oggi si apre una fase nuova e delicatissima del Paese, nel quale sono banditi i fischietti e gli spettacoli indecorosi, che qui dentro abbiamo visto, ma sono anche banditi i facili trionfalismi che abbiamo utilizzato in alcune fasi della gestione della pandemia. Come diceva il collega Errani, i dati della prima fase, che sono dati incoraggianti sulle vaccinazioni, riguardano il personale sanitario in una fase in cui le vaccinazioni alla popolazione non sono nemmeno iniziate. Possiamo concentrarci tutti, tutti, maggioranza e opposizione, sul lavoro da fare invece che sulla propaganda e la vendita di dati non ancora iniziati? Questo è fondamentale, senza accuse e senza critica. Mi rivolgo proprio al collega Errani: noi siamo pronti ad un lavoro di leale collaborazione. Ha fatto riferimento al piano vaccini, ai ristori e alle norme. Ministro, il primo terreno su cui creare collaborazione è il rispetto del Parlamento: mai più provvedimenti senza possibilità di discussione, abuso di DPCM, leggi di bilancio nemmeno aperte. Insieme alla collega Bonino, Operazione più Europa, abbiamo presentato una risoluzione, e io la ringrazio per l'attenzione che vi ha posto, che ha tre punti molto semplici: condivisione con le Camere del piano vaccini, trasparenza e comunicazione istituzionale, sorveglianza sulle proprietà immunologiche. Signor Presidente, ne approfitto per ritirare la premessa sulla quale il Governo non ha dato disponibilità e mantenere invece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

Senatrice Fedeli non riesce ad inserire la scheda? Non è collegato il *computer*?

dato che c'è stato qualche problema per la suddivisione dei vari senatori, per agevolare il computo dei voti, ai sensi dell'articolo 114 del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

ho deciso di intervenire oggi in Aula in quanto martedì, a Corato, intorno alle due di notte è stato appiccato un incendio dinanzi a una pizzeria. Sono al momento in corso le indagini per cercare di sapere chi sia il responsabile e per quale motivo sia stato compiuto tale gesto. Quello dell'altra notte è solo uno dei tanti eventi delittuosi che negli ultimi anni stanno avvenendo a Corato e nei paesi limitrofi. Una situazione insostenibile per la comunità. I dati rilevati dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, fanno emergere effettivamente un incremento dei reati consumati soprattutto per quanto riguarda i furti e i danneggiamenti,

di intervenire, e questa necessità è ancora più urgente oggi, in piena pandemia. Quindi, se da una parte è necessario sempre più l'intervento delle Forze armate, dall'altra, in considerazione dei concorsi espletati, chiediamo che sia assegnato personale appartenente alle Forze dell'ordine proprio a tutela dell'incolumità delle persone nonché delle attività imprenditoriali.

tra i quali 14 aree selezionate in Sardegna. Ferma la necessità, ormai urgente, di rendere pubblica questa mappa, al fine di avviare la complessa procedura di individuazione del sito più idoneo ad accogliere questi rifiuti radioattivi

ai costi che paghiamo in bolletta per conservare questi rifiuti, ma soprattutto ai problemi di sicurezza per le comunità che vivono negli attuali siti oramai precari. Nonostante ciò, però, non possiamo non ricordare ai nostri governanti quella che è la posizione politica e sociale dei sardi sulla questione. I sardi, già nel 2003, con una legge regionale si sono espressi formalmente sul divieto di impianti nucleari e sul divieto di stoccaggio di scorie radioattive nel territorio sardo, dichiarando la Sardegna territorio denuclearizzato. Ma c'è di più. Il popolo sardo, con un *referendum* consultivo, nel 2011 si è espresso in maniera quasi plebiscitaria (circa il 97,13 per cento) per il no al nucleare in Sardegna. allora, oggi il popolo sardo intende ribadire qui, in quest'Aula, in maniera ferma questa posizione, che vede tutti compatti, parti sociali e parti politiche, nel dire no al deposito delle scorie nucleari in Sardegna, nei 14 siti incomprensibilmente individuati dalla società Sogin. Questo perché lo stoccaggio in Sardegna comporterebbe problemi di trasporto in mare di materiale altamente radioattivo, perché la Sardegna ospita già importanti servitù militari (Quirra, Teulada, Capo Frasca), servitù industriali inquinate, aree mai bonificate che hanno danneggiato il tessuto agropastorale dell'isola. Penso a Porto Torres, al Sulcis. Non dimentichiamoci che la Sardegna è anche un'isola a vocazione turistica, con un patrimonio naturalistico, paesaggistico e archeologico da preservare anche da opere di questo tipo. Per questa ragione, come rappresentante delle istituzioni per i cittadini sardi, ribadisco con fermezza che tutto il popolo sardo, con la Regione e i Comuni capofila, presenterà al Governo adeguata e corposa documentazione scientifica atta a comprovare che la Sardegna non potrà mai essere sito per lo stoccaggio di scorie nucleari. Ringrazio tutta l'Assemblea. Presidente, colleghi senatori, le copiose nevicate che da Natale all'Epifania hanno interessato l'Appennino centro-settentrionale e l'arco alpino hanno provocato, ancora una volta, forti disagi e ingenti danni ai cittadini montanari. In particolare, sull'Appennino modenese non cadeva tanta neve dall'inverno 1985. Intere borgate sono rimaste isolate e senza corrente. Solo lo straordinario lavoro di privati e operai cantonieri ha consentito il transito sulle strade provinciali 324 e 486, nonché sulla statale 12 dell'Abetone. Tuttavia, a fronte degli oltre 2 metri di neve caduti ai passi dell'Abetone e delle Radici, i collegamenti con la Toscana hanno riaperto solo il 9 gennaio e ancora oggi il collegamento con la Garfagnana è chiuso causa slavine di neve, alberi e detriti. A vigili del fuoco, forestali, carabinieri sciatori, Protezione civile, agricoltori, operai provinciali dell'Enel e ai volontari tutti che hanno assistito le comunità isolate e stanno monitorando il rischio valanghe va il mio ringraziamento. Ora siamo però alla conta dei danni. Numerose aziende hanno subito il cedimento dei tetti dei capannoni sotto l'immane peso della neve e - solo per citarne una - lo stabilimento della Ceramica Alta del Comune di Frassinoro ha avuto danneggiati quei macchinari che danno lavoro a oltre 30 famiglie. Che dire poi degli immensi costi della spalatura neve? La sola provincia di Modena in questo inizio di inverno ha speso 300.000 euro di spandimento sale e spalatura. A -5 gradi il sale serve a poco e allora viene sparso con ghiaino, che andrà poi a intaccare il manto stradale. Quali e quanti saranno i danni sulle strade questa primavera? Quali e quanti i fondi disponibili per Province e Comuni? Cosa dire, inoltre, della tragica situazione degli impianti sciistici dei nostri comprensori? Nel Governo ci si accapiglia per le poltrone, mentre l'intero comparto turistico della montagna è allo stremo. Parliamo di un'ampia filiera, che comprende maestri di sci, impiantisti, albergatori, commercianti, ristoratori, lavoratori stagionali, un settore che, solo nell'Appennino emiliano, coinvolge oltre 2.000 persone. Le Regioni montane hanno stimato un danno di 12 miliardi e ne servono subito 5 a fondo perduto. Faccio mie le preoccupazioni del presidente di Federfuni, Andrea Formento, e del presidente del comprensorio di Cimone, Luciano Magnani, sollecitando il Governo a fornire aiuti parametrati alle entrate degli ultimi anni. In assenza di un movimento turistico che garantisce lavoro per tutto l'indotto economico, gli abitanti della montagna cosa faranno? Dovremo forse migrare a fare i tagliaboschi come facevano i nostri nonni? Ricordiamoci che un eventuale recupero su una stagione persa non può avvenire immediatamente, ma, per forza di cose, è necessario aspettare la successiva stagione. Ricordiamoci, inoltre, che la montagna rappresenta un territorio in cui i costi, le difficoltà e le scomodità sono nettamente superiori agli altri. Bisogna sostenere una precisa, puntuale e tempestiva valutazione pratica e non teorica in ambito di aiuti economici, in modo da scongiurare la ormai più che temibile caduta dell'economia montana. Quando un'impresa chiude in montagna, purtroppo, essa non riaprirà mai più, ricordiamocelo. Gli imprenditori di montagna non sono solo operatori turistici, sono anche sono anche operatori politici, poiché hanno contatto diretto con le persone che amano la montagna, ma che dalla montagna hanno ancora molto da prendere. Scongiurare la morte del turismo montano e non rimanere immobili è il proposito della Lega.

Signor Presidente, ancora una volta mi vedo costretto a parlare di cinghiali e lupi. i cinghiali sono infetti e untori di peste suina. Il ministro Bellanova dice che sta abbozzando un decreto per la prevenzione mediante un piano organico di gestione e controllo: il solito monitoraggio. Sulla A26, vicino a Novara, qualche mese fa sono morti due giovani

Per me andavano portati direttamente al ristorante. A Roma entrano in un parco giochi e vengono abbattuti: complimenti al dirigente che ha deciso. Qualcuno voleva adottarli e non cito il nome, per carità di Patria. Ad Asti un cinghiale ferito ferisce a sua volta un passante. In qualche appuntamento partitico di questi ultimi tempi qualcuno ha detto che occorre usare il contraccettivo: bisogna vedere chi va ad apporlo materialmente. Un'interrogazione da un membro di quest'Assemblea dice che si sta cacciando il cinghiale, nonostante i divieti, parlando a nome di milioni di italiani. Voglio parlare a nome degli altri milioni di Italiani, che spero siano di più, al di là dei partiti. Torniamo in noi:

telecamere fisse di proprietari di case di Piemonte e Liguria, nel caso specifico). Occorre ridurre il numero esorbitante di esemplari: si parla di 2 milioni, ma, a mio avviso, sono molti di più.

fare piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classe di età (non so come si possa fare) e formare i cacciatori; questi, però, cacciatori devono poter sparare sempre: viva la caccia! Le guardie venatorie provinciali vanno raddoppiate di numero, ma subito, perché il problema è vero e reale, per la sicurezza e l'incolumità delle persone. **Atti